la crisi storica che ha colpito il mondo occidentale, in particolare negli ultimi due anni, ha determinato la necessità di interventi strutturali nei processi decisionali dell'Unione europea. E infatti, come si è già avuto modo di discutere durante le valutazioni sulla Decisione di finanza pubblica circa 15 giorni or sono, sono stati previsti un nuovo meccanismo decisionale, l'introduzione del semestre europeo di bilancio, la rideterminazione del programma di stabilità e di crescita, che tiene conto di molte più variabili e, affiancato, il Piano nazionale di riforma *(National* *Reform Programme)*, che discutiamo nella giornata di oggi come progetto.

Sono nuovi documenti che nell'ambito europeo, ma a questo punto nell'ambito delle politiche nazionali, centralità politica assoluta e assorbente, come era stato dichiarato nel momento della Decisione di finanza pubblica. Con la crisi è nato quindi un nuovo disegno delle politiche europee, con la formalizzazione di tre processi. Un primo processo ha riguardato la riforma del sistema finanziario e bancario, al quale si affianca anche il percorso del cosiddetto accordo

Un meccanismo di sorveglianza macreconomica, quindi, con un monitoraggio degli squilibri strutturali delle varie economie europee. La severa sorveglianza, le sanzioni e il monitoraggio delle tendenze economiche e sociali sono vincoli ai Governi dei vari Paesi per le loro azioni; arriviamo alla stabilità dei conti pubblici, che diventa presupposto imprescindibile per la crescita, peraltro con la constatazione che non vi può essere crescita finanziata dai deficit pubblici.

che riesce a tenere il passo rispetto alle economie dell'Europa più avanzate, in particolare della locomotiva Germania, e un Sud senza un modello di successo); con l'indicazione delle politiche di agire, e quindi della necessità di interventi che abbiano valenza di regia nazionale; con la concentrazione delle risorse, in particolare quelle strutturali, sulle grandi infrastrutture; con un meccanismo di intervento sull'economia basato su aiuti sotto forma di fiscalità di vantaggio (venga prodotto il reddito e sarà detassato),

dirette) ad un modello federale, nell'ottica della nuova organizzazione dello Stato, e ad un sistema basato sui beni e sui consumi, anziché sui redditi e sulla persona. Il terzo obiettivo è una risposta alle difficoltà energetiche del Paese (quindi, la scelta nucleare). Si è competitivi se i fattori produttivi - e l'energia è un fattore produttivo fondamentale hanno prezzi competitivi, se vi è congruità rispetto agli altri Paesi concorrenti, e in questo momento per l'Italia così non è: in Francia l'energia costa la metà. Il quarto obiettivo è quello legale, è quello legale, su cui insistono i principi fondamentali di libertà. Il detto "tutto è libero tranne ciò che è vietato" non è ancora applicabile al nostro Paese,

Ostacoli che non si superano solo attraverso il controllo del debito pubblico, impedendone la crescita per favorire il rientro dal deficit.

di essere competitivi, con un mercato più aperto alla concorrenza, attraverso salvaguardie sociali che non siano rendite di posizione. colleghi, quante volte l'opposizione al cambiamento si è manifestata non sul merito, ma solo a difesa dell'esistente? I servizi pubblici devono essere efficienti ed efficaci e non necessariamente gestiti dal pubblico. Questi i grandi orientamenti, e al riguardo molto è stato già avviato. nella proposta, che la riforma pensionistica ci rende tra i migliori d'Europa in questo settore; che la riorganizzazione del nostro Stato secondo il modello federale ha l'obiettivo di compiere un passo in avanti anche nel

la privatizzazione con concorrenza in settori importanti, quali acque, trasporti e rifiuti. Il Programma descrive le fondamentali misure strutturali che, peraltro, sono parte integrante del programma di Governo

all'intervento nel mondo del lavoro teso a favorire - continuando sulla strada intrapresa - sistemi di contrattazione salariale e andamenti del costo del lavoro coerenti con la stabilità dei prezzi e capaci di promuovere la produttività. Anche su questo fronte molti passi in avanti sono stati compiuti, a partire dal modello del 2009, quindi dal modello di contrattazione, sia per la sua azione anti inflattiva (con l'esclusione del costo energia) sia, e fondamentalmente, sotto l'aspetto della contrattazione decentrata.

davvero convenire tutti sulla necessità di intervenire. sia nella burocrazia che grava sulle imprese. Questa è una strada già intrapresa con diversi provvedimenti, dalla direttiva sui servizi del mercato interno al decreto‑legge n. 78 del 2008, convertito nella legge n. 133, e alla legge di semplificazione attualmente *in itinere* in questo ramo del Parlamento. Sempre sullo stesso tema, vorrei ricordare le azioni relative al nuovo piano di logistica, che prevede lo sportello unico doganale, la riforma dell'autorità portuale, l'intermodalità e molti altri interventi. Ma ancora - e vengono richiamate nel Programma - le riforme dell'istruzione e dell'università, con un riallineamento alla media europea del rapporto insegnante-studenti, il superamento della disparità territoriale e un piano per la scuola digitale. Colleghi, ridurre l'abbandono scolastico La crescita dell'occupazione è favorita dalla coerenza del sistema della formazione e dell'istruzione con il mercato del lavoro,

del Programma riguarda l'ambiente e l'energia. Il documento prende in considerazione gli obiettivi che impegnano l'Italia a ridurre le emissioni secondo il Protocollo di Kyoto. In tale ottica,

Da ciò discendono le scelte di rifinanziamento dei fondi rotativi specifici relativi a Kyoto e quelli relativi alle fonti rinnovabili, ma da ciò discende anche la scelta di portare il nostro Paese alla costruzione di centrali nucleari.

La non congruità del costo energetico è da annoverare infatti tra le principali difficoltà delle nostre imprese nella concorrenza internazionale, ma anche tra le difficoltà del quotidiano, perché il costo dell'energia è un peso per ogni famiglia.

per una diversificazione produttiva di molte imprese: questo è affrancare l'Italia dalle servitù energetiche, oltre che uno stimolo alla ricerca, all'innovazione e a qualcosa di più moderno. Ricordiamo che la struttura del nostro sistema di imprese,

La combinazione tra imprese e organizzazione di centri pubblici rende dunque necessario prevedere sistemi di rete,

Le azioni si sostanziano, nell'immediato, nel rifinanziamento dei fondi esistenti per l'attuazione del Piano nazionale di ricerca e in una politica fiscale che incentivi i raggruppamenti di imprese a partecipare e a trasferire le conoscenze tecnologiche: l'innovazione di processo e di prodotto, non solo tecnologica - voglio ricordare, infatti, che l'Italia è anche il Paese della moda, dei grandi *brand* - è veicolo principale di sviluppo per il nostro Paese. L'ultima considerazione è legata al richiamo che all'inizio avevo fatto al dualismo nazionale Nord-Sud e alla capacità di spesa e gestione dei fondi comunitari. Si ribadisce che le risorse devono essere concentrate su grandi operazioni strategiche nell'ottica dell'obiettivo di Lisbona, e ciò deve valere sia per i fondi strutturali, i FESR, sia per la quota destinata al sociale, l'ex Fondo sociale europeo. La disponibilità di fondi per il prossimo triennio del programma 2007-2013

il Governo, per usare le parole del famoso libro del Ministro dell'economia («La paura e la speranza»), paralizzato dalla paura determinata dalle sue interne contraddizioni ed ormai sostanzialmente privo di speranza, sta facendo ogni sforzo per nasconderle al Paese, ma le novità che emergono dall'Unione europea per definire regole, sedi ed obiettivi del governo dell'economia a dimensione continentale sono davvero molto un Patto di stabilità e crescita - di questo si tratta - del tutto nuovo, orientato al superamento non solo degli squilibri delle pubbliche finanze, così come è stato fino a ieri, ma dell'economia reale ma dell'economia reale nel suo complesso. Le parole chiave, quindi, del nuovo Patto di stabilità e di crescita insieme a deficit e debito

bilancia commerciale, produttività, coesione sociale, lotta alla povertà, i dati della società e dell'economia reale. una novità sconvolgente, a fronte della quale la bozza di Programma nazionale di riforma di cui si sta discutendo questa mattina

la prima scelta nel processo di decisione del cosiddetto semestre europeo. Ecco l'altra enorme novità introdotta alla dimensione europea, in base alla quale le decisioni di bilancio e di politica economica, che verranno prese nella seconda parte dell'anno a partire dal 2011, saranno prese sulla scorta delle decisioni assunte nel semestre europeo. In sostanza, siamo di fronte alla sessione di bilancio dell'Unione europea. Cambia, di fronte a noi e in modo radicale, la realtà della gestione della politica economica e sociale. Il Programma nazionale di di riforma è una scelta ad altissimo contenuto politico, giacché si tratta di delineare puntuali obiettivi, quantitativamente definiti e dunque verificabili nel tempo, cui cui ispirare riforme strutturali volte al superamento dei cosiddetti colli di bottiglia, per usare l'espressione utilizzata nel documento della *task force* del Consiglio europeo, che restringono le potenzialità di crescita dell'Europa nel suo complesso e del nostro Paese. Proviamo dunque ad entrare nel merito, prima individuando le esigenze del Paese e poi confrontandole con la bozza che il Governo ci ha presentato. Lo farò mi scuso con i colleghi per la schematicità - ragionando per punti, un po' per esigenze di tempo, che è poco, un po' per fissare meglio i giudizi e le proposte essenziali.

la spesa pubblica, che nel 2009 ha raggiunto ben il 52 per cento del prodotto interno lordo, appena scalfisce il livello di disuguaglianza che si può calcolare prima dell'intervento dello Stato. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi

Peccato che, misurato il livello di disuguaglianza (cioè un indicatore di opportunità) prima dell'intervento pubblico e dopo l'intervento pubblico, risulta che in Italia si registra una riduzione, la quale però non è paragonabile a quella che si ottiene negli altri Paesi europei attraverso livelli di intervento pubblico nell'economia praticamente analoghi a quelli che si realizzano la mobilità sociale si è arrestata. La Banca d'Italia, in uno studio - non a caso, secondo me, completamente trascurato dalla politica italiana - ha dimostrato che, nel determinare il successo di un giovane, il luogo di nascita e le caratteristiche dei genitori continuano a pesare molto di più delle caratteristiche personali, come ad esempio il livello di istruzione acquisito.

secondo punto. La politica di consolidamento dei conti pubblici nel breve periodo determina inevitabilmente una minore crescita.

ma nel breve periodo le manovre di consolidamento dei conti pubblici, pur necessarie, determinano - ripeto - una riduzione della crescita.

per avere più crescita e più eguaglianza bisogna ridurre il debito, ma nell'immediato se si riduce il debito vi è una crescita minore di quella che avremmo se non lo facessimo. Questo è il circolo vizioso nel quale stiamo avvoltolati da molto tempo.

La prima è che bisogna realizzare una vera e propria rivoluzione nella qualità della spesa pubblica per renderla più produttiva sia in termini di efficienza economica, sia in termini di eguaglianza, mentre la si stabilizza prima e la si riduce poi, visto che - ripeto - la spesa pubblica ha raggiunto il 52 per cento del prodotto interno lordo e la spesa corrente primaria negli ultimi 10 anni è aumentata del 4,6 per cento ogni anno rispetto all'anno precedente. nel fatto che bisogna riconoscere priorità immediatamente a riforme che accrescano la produttività, ma non costano nell'immediato all'Erario; e queste riforme ci sono. Quinto punto. Il Programma nazionale di riforma deve avere, dunque, questa ispirazione e deve organizzarsi attorno a questi due obiettivi. Sul lato della finanza pubblica, la ristrutturazione deve riguardare sia il lato della spesa sia il lato delle entrate. Per il resto, le riforme devono interessare profondamente, se vogliamo aumentare la produttività

Quindi, le riforme devono riguardare i mercati dei fattori che, tradotto in linguaggio comprensibile, vuol dire lavoro, mercato del lavoro, energia, formazione del capitale umano, concorrenza nel cruciale settore dei servizi professionali, il in considerazione del fatto che il cattivo funzionamento di questi mercati è alla base della scarsa competitività del nostro sistema. Ecco, dunque, le riforme capaci di sciogliere il nodo della insufficiente competitività e della inaccettabile disuguaglianza che caratterizza il nostro sistema. Vorrei insistere su un punto che riguarda la perdita di produttività. Tra il 1998 e il 2008 il costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato del 24 per cento in Italia, del 15

naturalmente mi sto riferendo al settore privato. Poiché i salari in questi Paesi non sono aumentati molto da nessuna parte, se il costo del lavoro per unità di prodotto ha avuto tale andamento c'è una sola spiegazione: questo dato riflette una caduta drammatica della produttività del lavoro in Italia. Infatti, le cose sono andate in questa maniera: negli stessi anni la produttività del lavoro in Italia è aumentata del 3 per cento, in Germania del 22 per cento e in Francia del 18

marcati e persistenti dualismi - ecco la ragione - nella dimensione delle imprese e del mercato del lavoro.

comparto delle imprese produttive del settore manifatturiero che si sono ristrutturate e hanno fatto sacrifici drammatici. I lavoratori e gli imprenditori hanno investito ed innovato e sono diventati

non sono chiamate a reggere la competizione e quindi vivono con livelli di produttività assolutamente bassi, e non c'è mobilità tra questi due fattori. questi due fattori. Il dualismo del mercato del lavoro è l'elemento dominante del mercato del lavoro italiano, e strategie di unificazione sono note, non è che non non sappiamo come si faccia a procedere all'unificazione del mercato del lavoro: il fatto è che non abbiamo la forza, la politica non ha la forza di introdurre le innovazioni necessarie per affrontare questo tema e il dualismo del mercato del lavoro affossa le capacità competitive del sistema, oltre a provocare quella tragica ineguaglianza e ingiustizia sociale che ben conosciamo. Per i servizi, per i servizi professionali, per le attività dei servizi in rete come il gas, come il gas, da anni, dopo la parentesi brevissima, e non particolarmente incisiva, dei decreti Bersani, abbiamo interrotto il processo di liberalizzazione stiamo determinando buchi nella bilancia commerciale perché non siamo in grado di introdurre riforme che non costano in queste attività di servizio, che per noi, che siamo un Paese manifatturiero, sono essenziali per fare in modo che la nostra manifattura regga la competizione globale. Abbiamo quindi bassi investimenti in settori ad alta produttività, bassa spesa in ricerca, scarsa concorrenza: tutte cause generali che specificamente possono essere affrontate con singole riforme che non facciamo e, quindi, accompagniamo, come politica, il Paese nel suo declino. La sostanza è che su questo punto abbiamo bisogno di una sferzata meritocratica, di competizione e di apertura, ma in Italia, nel settore pubblico, le carriere e la crescita salariale avvengono solo per anzianità. Pensiamo al settore decisivo dell'istruzione e a quello della giustizia, alla magistratura: promozioni e salari crescono e si determinano solo per anzianità. Ma dove pensiamo di poter andare se il problema, nella società della conoscenza, è competere globalmente? settore privato abbiamo un presidio castale degli ingressi nelle attività da parte degli *insider* contro gli *outsider.* Ecco le riforme che non costano di cui c'è bisogno (l'elenco è naturalmente più lungo, ma avendo poco tempo, devo terminare).

la domanda politica sulla capacità del Governo di elaborare prima e guidare poi la realizzazione di un progetto che abbia questa ambizione. Conosciamo tutti la risposta a questa domanda: no, il Governo Berlusconi, anche ammesso che perduri la sua preagonica resistenza, è inabile allo scopo, non è in grado di realizzare questa strategia, nemmeno di elaborarla, come abbiamo visto dal documento. Nella coincidenza tra la formalizzazione della crisi del Governo e i giorni della presentazione del Programma nazionale di riforme è, direi quasi, icasticamente rappresentato il dramma del Paese: l'Italia l'Italia è obbligata a cambiare per non declinare ma è incapace di farlo per *default* della politica, cioè il soggetto regista e motore del cambiamento possibile. È per queste ragioni che abbiamo la necessità di sviluppare in queste ore qui al Senato un dibattito che ponga la crisi di Governo in atto sulle gambe di una valutazione dei problemi del Paese delle soluzioni da dare. Noi ne abbiamo presentate, nel corso delle discussioni dell'ultimo mese, di molto puntuali e precise, ma abbiamo di fronte un Governo che non c'è, che non interloquisce con l'opposizione su questo punto per la semplice ragione che il Governo da molto tempo non c'è più: c'è Tremonti. C'è il Ministro dell'economia, che nelle sedi europee,

ma è del tutto evidente che non è dentro questo processo. La signora Merkel, in un Paese di pochi abitanti e di scarso rilievo economico, è stata sette ore al *Bundestag* a rispondere alle osservazioni di maggioranza e di opposizione sul Consiglio europeo conclusosi la scorsa settimana con decisioni di portata epocale. In Italia, con tutto il rispetto per i Sottosegretari per l'economia che si susseguono a queste discussioni, noi abbiamo di fronte una tragedia. Il Presidente del Consiglio si occupa dei problemi che conosciamo bene, purtroppo, e il Ministro dell'economia, forse impegnato in queste riunioni europee, non trova nemmeno un minuto per venire a spiegare cosa diavolo stia facendo. Il problema è che il Paese ha bisogno di governo. Se voi non siete in grado di garantirlo, prendetene atto, dimettetevi subito e diamo luogo ad un confronto tra forze responsabili sugli interessi del Paese, per fare in modo che il Programma nazionale di riforma, di qui ad aprile, sia elaborato da un Governo capace di fare il suo mestiere.

della incapacità del Governo di assicurare al Paese la vitalità necessaria ad affrontare i difficili nodi che stanno di fronte a noi, questa prova sarebbe fornita, ed è fornita, dal testo del Programma nazionale di riforma. Questo programma, come hanno ben ricordato sia il relatore di maggioranza che quello di minoranza, non è un vuoto esercizio collocato tra la burocrazia e la retorica. È un elemento fondamentale della nuova *governance* europea che cammina su queste due gambe: un rinnovato programma di stabilità, in cui gli aspetti finanziari sono sottolineati con ulteriore vigore (debito e indebitamento) ma anche un'azione molto più incisiva per correggere gli squilibri strutturali delle economie europee, proprio attraverso questo strumento, il Programma nazionale di riforma, inserito pienamente nella procedura del semestre europeo. Programma che sarà esaminato dalla Commissione, la quale adotterà delle proposte di indirizzo che dovranno essere recepite nel bilancio degli Stati. I bilanci dei singoli Stati dovranno contenere le motivazioni e un giudizio sul grado di attuazione dei suggerimenti della Commissione. Dunque, si tratta di un documento e di un processo impegnativo. Per noi, poi, è particolarmente impegnativo perché, essendo più debole la situazione della finanza pubblica, siamo fuori

non cresciamo più. Cresciamo troppo poco. E la bassa crescita genera uno *stress* ulteriore della finanza pubblica e la pochissima elasticità della finanza pubblica impedisce politiche attive per correggere la bassa crescita. Dunque, dovremmo puntare, con molto più coraggio, ad introdurre quelle riforme a costo zero, o a basso costo, che possano correggere questo deficit

distacco, un'enorme perdita di prodotto. Tanto per fare un riferimento, ricordo che nella grande crisi, generata dallo *shock* petrolifero del 1974-1975, perdemmo il 3,8 per nella grande crisi finanziaria del 1992-1993 perdemmo l'1,9 per cento del PIL. È una crisi di dimensioni non conosciute e, nel frattempo, cambia la geopolitica.

del prodotto mondiale rispetto all'area dell'euro. Negli ultimi dieci anni abbiamo potuto contribuire alla crescita del PIL l'11 per cento con gli incrementi di produttività, mentre i nostri concorrenti europei sono cresciuti del 46 per cento. Solo un coraggioso piano di riforme può salvare l'Italia, e in questo progetto, signora Presidente, obiettivi numerici ambiziosi non sono sostenuti da politiche innovative; si parla di 2,2 milioni di poveri in meno, ma con quali politiche ciò si realizzerebbe, se avete azzerato il Fondo sociale e se non c'è alcun intervento per correggere la depressione dei redditi?

non si parla della riforma dei servizi. Fate una riforma una controriforma dell'avvocatura e scrivete nel Programma nazionale di riforma che il problema delle professioni è un problema che ritarda... la invito a concludere.

abbia dato significato al dibattito che dovremmo oggi sviluppare in quest'Aula. Credo altresì che il relatore di maggioranza si sia reso conto della distanza che separa tale documento dai provvedimenti che questo Governo e questa maggioranza hanno adottato e adottano in questo periodo di metà mandato. Lo scenario macroeconomico è complicatissimo; basta soffermarsi sul dato relativo agli investimenti fissi per il 2009, che segnala un meno 12

anno. Quindi in circa sei anni, dovremmo recuperare quanto è stato perso in termini di investimenti fissi nel corso del 2009. questo dato non riguarda soltanto il Mezzogiorno d'Italia, ma l'intero Paese. C'è addirittura una perfetta simmetria nella riduzione degli investimenti fissi, sottolinea la vanificazione dell'aggiuntività della spesa nel Mezzogiorno, finanziata dalle risorse comunitarie e segnala una situazione di grande difficoltà nella quale il Paese si trova ad operare. Quindi, non si capisce per quale ragione e sulla base di quali elementi si ritiene che il Nord del Paese rappresenti un modello di successo, che è equiparabile al modello tedesco e che quindi sostanzialmente non presenta problemi, quando invece il problema riguarda il nostro Paese. riguarda il nostro Paese in relazione anche agli obiettivi indicati al 2020. Voglio segnalare solo quello relativo

2,7 milioni di nuovi posti di lavoro in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Non mi pare che l'azione del Governo e le politiche in atto vadano in questa direzione. Ma, anche in questo caso, il divario maschi‑femmine in termini di occupazione, se presenta uno scarto di 30 punti nel Mezzogiorno, è rilevante anche nel resto del Paese. Nel Veneto quello scarto è pari a 22 punti,

tutto questo mentre sistematicamente vengono eluse le stesse decisioni che questa maggioranza aveva assunto con alcuni provvedimenti legislativi. legislativi. In questo progetto si cita la legge annuale per la concorrenza e per il mercato, legge che il Governo avrebbe dovuto presentare entro il 31 maggio, si ignora che la delega sulla riforma degli incentivi è stata sistematicamente spostata in avanti e si ignora anche che il programma operativo nazionale ricerca e competitività, che era dotato di 12 miliardi di euro, è stato ridotto a 6 miliardi di euro: di quei 6 miliardi, risultano spesi ad oggi meno di 700 milioni di euro, attraverso il meccanismo della rendicontazione di vecchi progetti realizzati con il decreto

che sono indispensabili per il Paese con l'azione quotidiana e con gli strumenti operativi che via via vengono approvati. *(IdV)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi. Libro dei sogni: già ieri, in occasione del dibattito che abbiamo svolto in Commissione finanze ho avuto occasione di esprimere - e non solo io, ma anche gli altri colleghi dell'opposizione - giudizi molto severi su un progetto di Programma nazionale di riforma se mi consente, signora Presidente - raffazzonato ed assemblato con una sorta di copia ed incolla. E non l'abbiamo detto solo noi ieri. Oggi, sulla prima pagina della «Repubblica»,

che non c'è più o che forse non c'è mai stato nel definire priorità e strategie di politica economica che andassero al di là del giorno per giorno», del tirare a campare, della palude dove si è inserito. Si tratta di documenti semplicemente incollati l'uno all'altro, senza neanche cercare di salvare le apparenze e mantenere le debite proporzioni. Questo non è un documento del Ministro dell'economia, è del Ministro delle politiche comunitarie, Ronchi, anche se il Ministro dell'economia, insieme al Presidente Berlusconi, qualche giorno fa, in conferenza stampa, ha difeso questo PNR.

in questi giorni «stanno finalizzando il vecchio programma nazionale di riforme basate sulla logica antecedente la discussione sulla riforma del Patto di stabilità. Siamo, tutti i Paesi d'Europa, al termine di una fase e al principio di una nuova». Per Tremonti si tratta di un documento importante, che ha definito "inventario di una serie di proposte", ossia la politica economica oggi si fa con gli inventari. Se passiamo ad esaminare questo documento, andiamo a vedere che altro che libro dei sogni! A pagina 11, quanto agli obiettivi al 2020 dell'Italia, il tasso di

I poveri invece stanno crescendo. Quindi chi sa in base a quale miracolo il Governo intende ridurre la povertà. Poi vi sono altre note squilibrate, anche negli indicatori principali fino al 2013, ossia il cambio dollaro-euro. Noi sappiamo che la valuta è in grande tensione in questi giorni e addirittura si fissa

la questione fiscale, il documento dedica una parte alla questione fiscale, alla riforma del sistema tributario con slogan, solo slogan assemblati e raffazzonati quando afferma che il sistema tributario prevede lo spostamento del peso dalla tassazione delle persone e dunque dai redditi personali alle cose, intese come consumo e proprietà, dalla complessità alla semplicità, dal centro alla periferia. Ma che cosa vuol dire tutto questo con una riforma fiscale che sarebbe necessaria per il Paese? Cosa vuol dire tutto questo con una armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie? Manca una armonizzazione delle rendite finanziarie. Voglio ricordare che il lavoro in Italia è tassato sopra il 20 per cento, al 22-23 per cento, e le rendite finanziarie sono tassate al 12,5 Manca anche questo. Mi faceva ricordare il senatore Pardi che in questo documento - ed è una beffa, soprattutto in un momento come questo in cui c'è il Veneto alluvionato, una Regione intera, e Vicenza è semidistrutta - manca del tutto il minimo di una politica ambientale e di difesa del territorio.

quella di ricordare in questo documento la "*farce action*" nella pubblica amministrazione, ossia la farsa dell'azione di classe nella pubblica amministrazione. Noi diamo un giudizio molto severo, signora Presidente, signori membri del Governo, su un documento che è solo un assemblaggio di buone intenzioni, che è slegato dalla realtà e che probabilmente rappresenta da parte del Governo gli ultimi giorni di Pompei.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la scelta compiuta dal Consiglio europeo di adottare la nuova Strategia «Europa 2020» dopo la grave crisi di questi anni consente finalmente di assumere unitariamente i due corni della vicenda dei singoli Stati, ovvero la necessità che i singoli Paesi adottino insieme due documenti strategici quali il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma. Insomma, il processo di risanamento della finanza pubblica, come nel nostro caso, deve necessariamente accompagnarsi a scelte volte a rilanciare lo sviluppo. Ci sono volute una importante scadenza imposta dall'Unione europea e la caparbietà dell'opposizione perché il Parlamento fosse chiamato a discutere di stabilità europea ed interna e di crescita e sviluppo, dopo una miriade di decreti-legge e di voti di fiducia che hanno scandito finora l'azione del Governo in materia di politica economica. Poteva essere una grande occasione di confronto e di condivisione per definire le priorità del sistema Italia, Paese riprenda a crescere superando antiche e nuove contraddizioni, ostacoli e ritardi, quelli che nel documento vengono chiamati colli di bottiglia. Così rischia di non poter essere, per un approccio burocratico e generico che il Governo ha adottato in questa così importante scadenza, nel disinteresse della propria maggioranza, o di quella che ne rimane in piedi, come vediamo in quest'Aula o come si è visto questa mattina in 14a Commissione, dove il parere della maggioranza è stato bocciato dai voti dell'opposizione. La scelta dei quattro obiettivi individuati verso cui orientare il Programma nazionale di riforma è una risposta parziale e insufficiente, pur richiamando titoli condivisibili ma dai contenuti assolutamente generici che dietro quei titoli si rivelano. in quel documento, pensate, proprio in questi giorni, quella che è da tempo una delle più grandi priorità del nostro Paese, cioè il suo dissesto idrogeologico, come dimostrato con sempre maggiore frequenza dalle continue tragedie che si verificano in prossimità dell'inverno; mi riferisco alle alluvioni, a quello che è avvenuto in questi giorni in Veneto e che sta avvenendo, probabilmente questa mattina, nel Salernitano. Parlate di Mezzogiorno ma replicate parole vuote, a cominciare dal fantomatico piano per il Sud, senza alcun concreto riferimento alle risorse saccheggiate in questi anni e a quelle che il Governo ha deciso di centralizzare e di cui tuttora non si intravede alcun concreto programma di impiego. Parlate di fiscalità ed esaltate il federalismo fiscale, che ad oggi è ancora per vostra responsabilità una scatola vuota, ad un anno e mezzo dall'approvazione della delega. Parlate di concorrenza, ma dimenticate di essere uno dei Governi che più di altri ha affossato le liberalizzazioni e le aperture ai mercati, ripristinando vecchie protezioni corporative, e che ha dimenticato nel cassetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza. Infine, parlate di energia, ma sostanzialmente per ribadire la scelta del nucleare, rinunciando ad affrontare con modernità e concretezza uno dei fattori decisivi per il futuro produttivo e sociale del Paese. Aver deciso di esaltare in modo così esasperato e con argomenti propagandistici e forzati la scelta del nucleare all'interno di questa bozza di Programma nazionale delle riforme, è davvero il segno di un'opzione ideologica più che di mercato e strategia. Una strategia, quella energetica nazionale, che, vorrei ricordare, ancora non è stata presentata dal Governo al Parlamento, anche qui ad un anno e mezzo dalla legge che prevedeva tale adempimento. Parliamo di uno strumento di programmazione che doveva anticipare e non certo seguire le scelte del Paese in materia di energia. Una solida e seria strategia energetica nazionale, più che brandire vessilli ideologici farebbe i conti, da un lato, con la consapevolezza della perdurante sofferenza del Paese verso un *mix* energetico oneroso, troppo dipendente dall'importazione di idrocarburi, e, dall'altro, con la grave crisi, che ha contribuito a modificare profondamente gli stessi scenari per la produzione e il consumo di energia sia per l'Italia, che per gli altri grandi Paesi europei per i prossimi anni.

L'Italia può giungere a quelle date, in primo luogo, rispettando e possibilmente migliorando l'obiettivo del 17 per cento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, allineandosi in tal modo ai principali Paesi europei, ottimizzando, in secondo luogo, la capacità produttiva delle centrali convenzionali (la cui potenza al 2020-2030 sarà in eccesso per via dell'attuale disponibilità di impianti, cui si aggiungeranno quelli in costruzione), in terzo luogo investendo con più coerenza e convinzione di quanto fatto finora su efficienza e risparmio energetico, la declinazione più significativa già da subito della strategia energetica nazionale. Fa specie Fa specie che, pur richiamato nella bozza di Programma nazionale di riforma, ad oggi, non vi sia alcuna certezza per i consumatori nonché per il sistema delle imprese del rifinanziamento della deduzione del 55 per cento delle spese per l'efficienza energetica in edilizia; un intervento che finora, in quattro anni, ha registrato nel nostro Paese 800.000 beneficiari e 11 miliardi di euro di investimenti; una iniziativa cruciale richiamata proprio in queste ore dal commissario europeo all'energia Oettinger, che ha annunciato per oggi una proposta effettiva per raggiungere al 2020 il 20 per cento di efficienza energetica in Europa. Così come non vi è traccia nella bozza di Programma nazionale di riforma della necessità di riprendere il processo di liberalizzazione del mercato energetico, a cominciare dal gas e dalla non più prorogabile vicenda di SNAM-Rete gas, così come chiedono da anni l'Europa e l'Autorità. Non vi è traccia infine dello sviluppo della tecnologia della cattura e del sequestro della CO2, cui l'Europa ci sollecita e che vede l'Italia in grado di produrre una tecnologia ampiamente esportabile in tutto il mondo, poiché poiché interessa un gran numero di Paesi, anziché metterci alla coda di altri Paesi con il vecchio nucleare, di cui noi disponiamo, né di tecnologia, né di materia prima, né di impianti di arricchimento dell'uranio, né di depositi per i rifiuti radioattivi; insomma, una scelta che aumenterebbe la dipendenza dell'Italia da altri Paesi e dalle importazioni, nonché una scelta particolarmente onerosa, al contrario di quanto da voi sostenuto. Un'occasione persa, insomma, questa bozza di Programma nazionale di riforma. Peccato!

Signora Presidente, penso che la discussione che stiamo sviluppando sul piano delle riforme avrebbe meritato non solo un'attenzione, ma anche una presenza del Governo adeguata.

il Ministro dell'economia è stato sensibilizzato ed ha partecipato ad una riunione delle Commissioni esteri di Camera e Senato, unitamente alle Commissioni bilancio, per rappresentare la linea che intendeva sostenere in seno a quella che sarebbe stata la prima riunione

cogliendo gli elementi di ricerca e di *governance* mondiale che erano stati posti all'attenzione della crisi.

l'Unione europea, il Ministro dell'economia italiano si è mosso come se fosse una sorta di governatore unico. Abbiamo per caso scoperto che nel mese di luglio ha depositato un documento contenente la valutazione che l'Italia faceva delle misure che dovevano essere adottate, documento che - come risulta da una rapida ricerca - non è stato discusso in nessuna sede. sede. Anche la discussione odierna, a partire dal dibattito che si è svolto non più tardi di una settimana fa in questa sede prima del Consiglio e che poi ha finito per svolgersi in contemporanea con l'ultimo Consiglio europeo,

senza che siano precedute da un approfondimento assolutamente proporzionato all'importanza delle decisioni? Ho provato a darmi una spiegazione. Una prima spiegazione convincente può essere che la crisi politica della maggioranza è talmente profonda,

di dare la sensazione che l'Italia non sia in grado, non solo di discutere, ma soprattutto di decidere. Quindi, ha ritenuto più opportuno decidere da solo.

sono solo indicate delle misure. A mio avviso, la discussione dovrebbe incentrarsi più sulla nota aggiuntiva che accompagna il documento che non sui contenuti, perché su quelle misure è difficile registrare

quest'Aula, trovandoci d'accordo sull'analisi per poi scoprire che vi erano delle differenze profonde squisitamente di opportunità politica nelle conclusioni. Basti pensare alla discussione che abbiamo fatto ogni volta che ci siamo soffermati su come governare la spesa e su come riportare sotto controllo la spesa del nostro bilancio. Tuttavia le quattro azioni indicate nella nota aggiuntiva nota aggiuntiva meriterebbero un'ulteriore discussione, un ulteriore approfondimento, perché non si intravede in quelle azioni, in ciascuna di esse, qual è la priorità che il Governo sceglie nell'arco del periodo temporale

dei meccanismi di coordinamento predisposti dall'Unione europea per il conseguimento, non soltanto della stabilità finanziaria pubblica - come si è tentato di fare fino ad oggi,

L'altra premessa fondamentale, com'è stato ricordato in alcuni interventi, è la nuova strategia adottata dal Consiglio europeo, che va sotto

nella mancanza di coordinamento delle politiche economiche e di riforma poste in atto dai diversi Stati a sostegno dell'obiettivo fondamentale. Europa 2020 è una Strategia nuova, che cambia gli obiettivi fondamentali, sostanzialmente integrando quello dell'economia della conoscenza - riassunta nella parola "*smart*" (la crescita intelligente) con altri due termini che erano rimasti un po' in ombra in quest'ultimo decennio, vale a dire la sostenibilità e l'inclusività della crescita.

in realtà è conseguenza anche del fatto di non riuscire più a realizzare quella competitività basata sulla qualità del capitale umano e del lavoro su cui si era puntato con la Strategia di Lisbona.

o ancora organizzativo-imprenditoriale. In realtà, la conoscenza, in particolare quella tecnico-scientifica, è ormai molto diffusa nel mondo e le eccellenze non sono più solo nei Paesi di più antica industrializzazione come l'Europa ed in parte anche in Italia. Da questo punto di vista bisognerebbe peraltro dire che si dovrebbe rafforzare di molto il nostro sistema formativo, poiché molte statistiche evidenziano la sua caduta rispetto agli standard internazionali. Il rischio purtroppo è anche un altro, ed è legato al fatto che la crisi degli anni 2008-2010

fatto andando ad incidere proprio sulla capacità di investire su quegli *asset* che vanno in direzione degli obiettivi di Europa 2020.

per il sostanziale fallimento della Strategia Europa 2020 su cui si dovrebbe reggere la competitività dei Paesi europei e anche dell'Italia negli anni a venire. Ecco perché questo Programma nazionale di riforma è davvero fondamentale per noi. Sappiamo che esso rappresenta in realtà il primo tentativo che l'architettura europea pone in essere per coordinare le politiche economiche e non più soltanto gli obiettivi di stabilità finanziaria pubblica, come era stato fino ad ora. Proprio per questo, partendo dalla bozza odierna, credo che il Governo e tutte le forze politiche debbano fare uno sforzo di riflessione molto importante per includere in questo Programma le riforme di le riforme di sistema, le riforme strutturali che incidono sui fattori produttivi che rendono maggiore o minore - e in questo periodo storico purtroppo non molto elevata - la nostra competitività sul piano internazionale.

- dal punto di vista della capacità produttiva e della qualità del fattore umano - intesa storicamente come capacità di apprendimento stratificate nella società, nei lavoratori e nell'imprenditoria del nostro Paese, sia alla crescita sostenibile, per le potenzialità che il nostro patrimonio ambientale, storico, artistico, culturale

posizioni a livello mondiale. Ora, rispetto agli obiettivi di Europa 2020 l'Italia non è messa male; però in questo Programma nazionale di riforma deve fare intravedere riforme strutturali, capaci di cambiare davvero le condizioni della competitività del Paese in questi settori e non semplicemente volte ad allocare le proprie politiche di spesa o addirittura ad allocare i fondi europei che saranno copiosamente, negli anni a venire, destinati al raggiungimento di questi obiettivi.

questo punto di vista, esso può scontare un difetto naturale legato anche alla grande tempestività con cui è stato predisposto e al fatto che su queste politiche si deve avviare un percorso di riflessione comune. È fondamentale però che da qui ad aprile tale percorso si

È veramente singolare che un documento di tal genere e di tal peso sia stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 novembre scorso, ben sapendo che esso doveva essere presentato in sede comunitaria nei primi giorni di novembre,

che nell'arco di un'ora una Commissione possa serenamente, onestamente ed in termini concreti esprimersi su un documento del genere, nel cui frontespizio

slancio alla nostra economia e a quella degli Stati membri. Infatti, il Programma nazionale di riforma si pone in linea di continuità con i piani per la crescita e l'occupazione già approvati nel 2005 e nel 2008 nell'ambito della Strategia di Lisbona. Appare però molto più stringente in quanto è stato procedimentalizzato l'*iter* (secondo quanto indicato nella nota aggiuntiva). Una delle critiche mosse infatti alla Strategia di Lisbona era quella della mancanza di una procedura che valesse a dare compiti e ruoli ai vari soggetti interessati, che si traduceva di fatto nella mancanza nei Governi degli Stati di stimoli all'effettuazione degli interventi previsti. È evidente che nel mondo globalizzato, le sfide che attendono i singoli Paesi Paesi dell'Unione europea vanno affrontate congiuntamente e in un'ottica sinergica tra dimensioni nazionali e dimensione comunitaria. Dall'intreccio delle competenze e delle risorse deve essere sospinto il rilancio dell'economia europea, in difficoltà rispetto non solo ai tradizionali competitori sulla scena internazionale, quali Stati Uniti, Giappone, Canada, ma anche rispetto a realtà quali la Cina, l'India e altri Paesi emergenti, venuti prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, grazie alla liberalizzazione

avendo assicurato ai Paesi dell'Unione una ricchezza e un benessere collettivo che, almeno sinora, ha rari eguali nel mondo. È dunque da accogliere con favore la espressa inclusione delle Camere nella procedura di adozione del Programma di riforma. L'obiettivo strategico che ci poniamo è raggiungere da qui al 2020 un livello minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, destinata alla ricerca e innovazione pari all' 1,53 per contro l'attuale 1,1 per cento. Per questo il Governo intende tra l'altro attuare il programma nazionale della ricerca così da «allineare la spesa italiana in questo settore alla media europea». L'elenco delle linee di azione che il Governo intende mettere in campo (variabile politica permettendo) è contenuto nella bozza del Programma nazionale di riforma, che è il primo degli adempimenti previsti dalla nuova *governance* economica europea. Il documento dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 12 novembre in versione preliminare, mentre l'integrale è atteso per il mese di aprile insieme all'aggiornamento del Programma di stabilità. Federalismo fiscale, riforma della tassazione, previdenza, competitività e riforma della pubblica amministrazione: è questo l'elenco delle misure in cantiere e degli effetti attesi dalle riforme già avviate. si può notare si tratta di nutrito programma. Lo scenario è costituito dagli obiettivi della Strategia Ue 2020 per la crescita e l'occupazione. l'occupazione. Sul fronte dell'energia, la strategia di lungo termine - si legge nel documento - «impone *hic et nunc* l'avvio della reintroduzione della produzione elettronucleare nel nostro Paese attraverso l'installazione di impianti a tecnologica nucleare di terza generazione avanzata». Circa 9 miliardi di fondi gestiti dalle Regioni saranno indirizzati all'efficienza energetica e al potenziamento dei servizi ambientali. Nel campo dei mercati energetici il Governo «procederà al recepimento delle direttive del cosiddetto terzo pacchetto mercato interno». Sulla scuola, gli obiettivi in tema di abbandoni vengono indicati con percentuali importanti. Per l'università, nel documento si indica come «obiettivo primario» l'eliminazione della frammentazione degli indirizzi, accanto al sostegno della qualità dell'offerta formativa. Gli investimenti totali dedicati all'istruzione vengono quantificati in circa 4,3 miliardi di euro, 3,8 dei quali sono destinati «ad azioni di riforma dei sistemi di istruzione e formazione, per sviluppare l'occupabilità e aumentarne la pertinenza rispetto alle esigenze del mercato del lavoro». Per quel che riguarda il mercato del lavoro, l'obiettivo 2020 si colloca in un intervallo tra il 67 e il 69 per cento per il tasso di occupazione. *Target* condizionato «dall'intensità della crescita», che potrebbe tradursi in un incremento dell'occupazione di 1,6-1,8 milioni di unità.

all'interno della strategia complessiva per l'occupazione «l'incremento del tasso di occupazione per le donne riveste un ruolo chiave». Per le politiche di inclusione sociale previste a livello comunitario, sono previste per l'intero decennio risorse per 3,9 miliardi. Per questo è necessario mettere in campo ogni utile iniziativa affinché le donne possano fornire il proprio contributo e ciò sarà possibile attraverso azioni mirate e integrate che ne aumentino il peso nella politica, nelle istituzioni, nel mondo del lavoro e in posizioni apicali. un ultimo passaggio per quanto riguarda un uso più efficiente delle risorse femminili nel mercato del lavoro ed una maggiore presenza di imprenditoria femminile, che possono favorire il conseguimento di un'economia sostenibile e giusta e più attenta alle esigenze dell'ambiente. Infatti, la *green economy* rappresenta la nuova frontiera su cui investire e attraverso la quale si apriranno nuove prospettive ed opportunità per moltissime donne. Tralascio il resto dell'intervento, che consegnerò. Sottolineo soltanto, in chiusura, l'importanza del Programma nazionale di riforma che, come ho detto, rappresenta una grande opportunità per dare slancio alla nostra economia e a quella degli Stati europei; tuttavia, vista la rilevanza degli argomenti trattati sarebbe stato necessario avere più tempo a disposizione del Parlamento per affrontare le innumerevoli tematiche; non esiste, infatti, alcun obbligo giuridico di trasmettere questo progetto alla Commissione europea entro il 12 novembre. La fretta con cui dobbiamo esaminarlo rischia purtroppo di rendere totalmente privo di forza un Programma, che nelle intenzioni deve rappresentare un contributo alla stabilità, alla crescita ed alla credibilità del nostro Paese nel sistema economico europeo.

ed in modo particolare del Mezzogiorno d'Italia, che credo sia assolutamente offensiva di questo Paese. Cito testualmente, così comprendiamo meglio di cosa stiamo parlando: nel Programma nazionale che ha la presunzione di chiamarsi «di riforma» e che mi sembra più un adempimento burocratico, per come il Governo lo sta affrontando e lo ha affrontato, e un po' indecente per come lo sta proponendo in Parlamento, al al capoverso che riguarda gli obiettivi da raggiungere pone quattro questioni essenziali e la prima è la cosiddetta questione meridionale. Non credo sinceramente che possa essere così rappresentato in Europa il nostro Paese, non tanto perché non vi siano elementi di realtà e verità nelle considerazioni che si possono fare su come questo Paese è cresciuto negli anni, quanto soprattutto per il modo con cui tale quadro può essere interpretato dagli operatori stranieri che nel nostro Paese sono chiamati ad investire. [**Presidenza si dice che «L'Italia è un Paese ad economia "duale". Non vogliamo che diventi un Paese diviso. Le statistiche nazionali, fatte su medie non mediane, non rappresentano adeguatamente questa realtà. Il Centro-Nord ha consolidato un elevato livello di sviluppo. Il punto è che il Centro-Nord ha già un modello di sviluppo di successo, che non è fondamentalmente diverso da quello tedesco. Il rafforzamento della sua competitività è un processo difficile e duro, poiché la distanza che ci separa dalla Germania è ancora tanta. Ma è un procedere nella continuità Per contro il Sud non ha un modello di sviluppo di successo e quindi il suo non può essere un processo nella continuità, ma basato sulla discontinuità. Rispetto allo sviluppo è un prerequisito la normalizzazione del territorio, attraverso la lotta alla criminalità». Mi fermo qui, perché voglio evitare di leggere ulteriori considerazioni che offenderebbero i colleghi qui presenti in Senato e anche la nostra intelligenza; ma è vergognoso

sede. Il fatto che siamo nella prima fase di esame di un modo nuovo di concepire la programmazione ed il dibattito parlamentare sulla programmazione economica e finanziaria - e quindi scontiamo anche i limiti di un tempo molto ristretto entro cui esaminare ed affrontare il Programma nazionale delle riforme, perché c'è la scadenza del 12 novembre di merito dei documenti. Si tratta infatti di documenti che vengono poi consacrati da atti parlamentari e che diventano l'oggetto di una trattativa e di una piattaforma di discussione in sede europea, in cui il nostro Paese si qualifica per le riforme che intende attuare. Non è accettabile, signor Presidente, che si dia una rappresentazione di questo Paese in cui è sconsigliato e sconsigliabile investire nel Mezzogiorno d'Italia, perché ha un'economia prevalentemente sottosviluppata e criminale. Criminale è questo modo di interpretare i problemi del Paese: non è accettabile, da parte di nessuno. A ciò voglio associare anche lo scandalo di un modo di procedere nell'esame del Programma nazionale di riforma, in Commissione bilancio e nelle Commissioni di merito, in contemporanea, oggi, con la discussione generale dello stesso Programma di riforma,

che, francamente, non è accettabile questo modo di procedere sui conti pubblici, sulle scelte di riforma economica e sociale riguardanti questo Paese, sul modo di affrontare la crisi la crisi e di rappresentare un modello virtuoso che non c'è, perché questo modello virtuoso, purtroppo, annega nelle alluvioni di questi giorni, che rivelano le inefficienze di un sistema infrastrutturale, esistenti al Nord, al Centro e al Sud di questo Paese. Questo modo vergognoso di rappresentare il nostro Paese non solo non ci sta bene, ma dovrebbe far indignare più di qualcuno e dovrebbe anche farci individuare un modo più serio di affrontare questioni strategiche riguardanti le riforme economiche di questo Paese. Signor Presidente,

Quindi, io pongo una questione di metodo e una di merito, che ci pongono, veramente e scandalosamente, in una condizione disarmata rispetto a chi se ne "strafrega" di quanto sta accadendo in questo Paese.

io credo che l'inadeguatezza di questa bozza di Programma di riforma sia dimostrata già soltanto dalla distanza esistente tra i titoli dei vari capitoli e il modo in cui questi titoli vengono sviluppati. Uno dei cinque temi nella bozza, come oggetto della cosiddetta sorveglianza, è quello che viene definito economia ecoefficiente e cambiamenti climatici. all'interno di questo capitolo più di metà dello spazio è assorbito dal cosiddetto programma nucleare del Governo.

per ragioni di sicurezza; per ragioni di accettabilità sociale; per il modo in cui è stata organizzata la *governance* intorno a questo programma. Però, anche lasciando da parte questa nostra posizione, il programma nucleare non ha davvero nulla a che fare né con l'economia ecoefficiente, né con i cambiamenti climatici. Non ha nulla a che vedere con l'ecologia, e mi sembra persino superfluo spiegare il perché, e non c'entra assolutamente nulla con l'efficienza energetica. Si può essere a favore o contro l'energia nucleare, ma nessuno che abbia anche i minimi rudimenti di ingegneria potrà mai sostenere che passare da una centrale tradizionale a una nucleare faccia guadagnare qualcosa in termini di efficienza energetica nella generazione o nei consumi non c'entra nulla con i cambiamenti climatici, che sono oggi legati a tre obiettivi che hanno come scadenza il 2020; meno 20 per cento di consumi energetici, cento di emissioni clima alteranti, più 20 per cento di fonti rinnovabili. Ebbene, credo che nessuno, nemmeno il più fanatico dei fautori del nucleare, può sostenere che realisticamente nel 2020 in Italia saranno già entrate in funzione

Le enunciazioni sono in parte condivisibili, anche se un po' meno condivisibile è la premessa per cui l'Italia, dal punto di vista dell'efficienza energetica, sarebbe all'avanguardia in Europa: infatti, l'unico campo e settore dove questo è vero è quello della generazione elettrica, ma nel campo dei trasporti, come nel campo dei consumi civili e residenziali, l'Italia è drammaticamente indietro rispetto agli altri principali e più avanzati Paesi europei. Si dice poi correttamente che una delle misure più promettenti e che hanno dato risultati migliori in questi anni dal punto di vista del miglioramento dell'efficienza energetica (proprio in uno dei settori più critici, quello dei consumi è il cosiddetto credito d'imposta del 55 per cento concernente le ristrutturazioni energetiche. Già il senatore Tomaselli ha ricordato alcuni dati di bilancio di questi quattro anni di applicazione dei cosiddetti incentivi del 55 per cento: sono stati aperti più di 800.000 piccoli cantieri, che vuol dire che 800.000 e più famiglie o condomini hanno deciso di intervenire e di spendere dei quattrini per migliorare il rendimento energetico delle loro abitazioni e dei loro palazzi, perché c'era e c'è l'incentivo del 55 per cento. Il mercato che si è creato grazie a questa misura dal punto

Vorrei ricordare che il 31 dicembre di quest'anno il credito d'imposta del 55 per cento scade: non si sa se, *in extremis*, in «zona Cesarini», il Governo deciderà di prorogarlo, ma ciò che è certo è che da alcuni mesi questo mercato è fermo. Infatti, nessuna famiglia e nessun condominio decidono, nell'incertezza della prosecuzione degli incentivi, di realizzare questi interventi. Credo quindi che, al di là

provvedendo a stabilizzare una misura che ha dato buoni risultati da tutti i punti di vista. Credo che sempre di più questo Governo e questa maggioranza dimostrano un'incapacità di passare dalle parole ai fatti - persino dalle loro parole ai loro fatti - e mi pare che questa bozza di Programma nazionale di riforma sia la fotografia più fedele di questo collasso.

elaborata dalla Commissione europea nel marzo di quest'anno. Questa strategia, che sostituisce la precedente Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione - che, obiettivamente, presentava dei *goal* che non sono stati centrati, forse anche perché troppo ambiziosi - integra anche le procedure relative alla stabilità dei conti pubblici degli Stati membri nell'ambito del nuovo semestre europeo, che prevede a partire dal 2011 la presentazione del Programma nazionale di riforma e del Programma di stabilità. La scelta iniziale di un'Europa solo funzionale sta poco a poco cambiando, non è più sufficiente, è stata superata dalla situazione contingente: la crisi globale che ha colpito il pianeta ha portato inevitabilmente a questo. Un'area così grande, che vuole veramente contare, deve essere organizzata in modo più omogeneo anche dal punto di vista economico-finanziario. Proprio con la legge comunitaria 2009 è stata introdotta, all'articolo 4-*ter*, la norma in base alla quale il Governo è tenuto a consultare e informare le Camere nella predisposizione del piano nazionale di riforma, nonché a trasmettere la bozza prima della presentazione alla Commissione europea per l'adozione di eventuali atti di indirizzo.

Ricordo, per chi non se ne fosse mai accorto, che negli anni precedenti non si parlava di piano nazionale di riforma, ma si parlava di PICO, che era più o meno la stessa cosa. Il Programma analizza in modo approfondito lo scenario macroeconomico e i principali squilibri del sistema italiano, sistema che presenta alcune criticità, prima fra tutte il debito pubblico, che rappresenta un vincolo non eludibile per qualunque tipo di analisi e qualunque tipo di obiettivo si voglia raggiungere. Nel documento viene ben evidenziato che non esiste crescita senza stabilità dei conti pubblici. Non si può pensare di crescere incrementando il deficit pubblico; questo deve essere molto chiaro per tutti e deve essere alla base di ogni proposta legislativa per lo sviluppo. Credo che la finanziaria triennale adottata all'inizio di questa legislatura vada esattamente in questo senso, così come va in questo senso la riforma del sistema pensionistico, che, partita nel 1995, con successivi ritocchi fino all'ultima decisione del luglio scorso, ha dato una grande iniezione di stabilità ai conti del Paese. Ma per crescere il nostro Paese ha bisogno di sciogliere anche altri nodi (come evidenzia appunto il documento), quali lo sviluppo del Meridione, un ammodernamento del sistema fiscale trovare le condizioni per produrre energia a costi più bassi. Sappiamo che il costo dell'energia è uno degli handicap più grossi per la competitività delle nostre aziende; credo quindi che

il sistema giustizia, che, per quanto riguarda la giustizia civile, va sicuramente ammodernato: ci sono infatti troppe lungaggini e troppe regole. Il documento, come dicevo, individua i principali squilibri del sistema italiano: oltre al debito pubblico, le carenze di competitività, di produttività, consistenza ed efficienza amministrativa, di conoscenza, di ricerca, la necessità

lo sviluppo del Sud e il federalismo fiscale, che sono, a mio parere, due facce della stessa medaglia. Il modello di sviluppo del Sud va cambiato. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che non è dando più soldi e più fondi che si sviluppano quei territori. Questo è stato fatto nel passato e non mi pare che sia servito a molto. Si è parlato molto di fondi comunitari; io parlerei, effettivamente, di perdita di un'occasione con la perdita della capacità

che non hanno lasciato nulla per quello che riguarda lo sviluppo del territorio. Non solo. Risulta - recentemente la Corte dei conti ha tenuto su questo un seminario - che gran parte dei fondi nazionali ed europei,

Si parla del 70 per cento, e all'interno di questo, il 30 per cento solo in Calabria. Immaginate che cosa avrebbe potuto rappresentare per lo sviluppo di quelle Regioni l'uso corretto di quei fondi comunitari. Adesso ne arriverà un'altra fetta e io credo che sia fondamentale intanto aiutare queste Regioni a fare dei progetti per spenderli, perché purtroppo sono un pochino carenti. Da questo punto di vista, quindi, forse una cabina di regia regia sovraregionale è assolutamente necessaria: hanno infatti dimostrato che da soli lì non ce la fanno. E poi, importantissima, rispetto a quello che dicevo sulle frodi, è una normalizzazione del territorio attraverso la lotta alla criminalità, cosa che mi pare questo Governo stia facendo in modo molto serio. Il ministro Maroni insieme alle forze della magistratura, a tutte le forze di polizia, sta lavorando molto su questo. Altrimenti, tutti i soldi che diamo finiscono, invece che in progetti di sviluppo, nelle tasche di qualcuno che non si merita di averli. Il vero Il vero sviluppo del Sud, quindi, passa attraverso un uso oculato di questi fondi (e anche nel programma 2007-2013 vi è ancora una bella fetta che dobbiamo spendere) e poi attraverso crediti d'imposta, fiscalità di vantaggio: tutte cose che comunque questo Governo ha messo in agenda. L'altro versante, il federalismo fiscale, ha iniziato il suo cammino lo scorso anno e sta andando avanti: vedi il decreto sul federalismo demaniale, adesso quello sui fabbisogni e costi standard, che ci auguriamo al più presto possa essere licenziato anche dalla Commissione paritetica con un parere favorevole. favorevole. Io credo che in un sistema a tutti gli effetti di sviluppo duale, come è quello italiano, il federalismo sia assolutamente indispensabile perché rappresenta l'unico sistema in in grado non solo di tenere insieme il Paese ma di permettere ricette di sviluppo differenziate a seconda delle esigenze dei territori. È quindi fondamentale. Certo,

Ashton, in seguito alle calamità naturali in Pakistan, si è deciso di non dare più fondi ma azzerarli riguardo al tessile. La valutazione di Gianfranco Dell'Alba è la perdita, solo in Italia, di 30.000 posti di lavoro. Questa informazione forse è sfuggita!

porta la firma del ministro per le politiche europee Ronchi, per cui mi sarei aspettata che, insieme ai Sottosegretari all'economia, il ministro Ronchi, che è stato quello che ha coordinato il lavoro, venisse a sentire che cosa ne pensa questa Assemblea del Senato. Ci sarebbero moltissime altre cose da aggiungere; mi limito ad una. La Commissione politiche dell'Unione europea

frontespizio del documento si fa riferimento ad una bozza che il Governo si è impegnato ad inviare all'Unione europea entro l'autunno 2010. Il documento finale sarà spedito nell'aprile 2011 e, quindi, io assumo che l'esame di quest'oggi sia l'avvio di una discussione che si completerà nell'aprile del prossimo anno. Nel dire questo, ricordo, in in quanto da tanti anni in Parlamento e con un recupero di memoria, che è la terza volta nella storia del nostro Parlamento che si discute e si affronta un documento di pianificazione avente un arco temporale di dieci anni: la prima volta fu all'inizio degli anni '80, con l'esperienza dei primi Governi di centrosinistra;

sono contenute riflessioni e affermazioni straordinariamente importanti che credo anche i colleghi della minoranza non dovrebbero sottovalutare e se convenissero con noi

la crisi finanziaria che ha sconvolto l'intero mondo occidentale ha imposto un nuovo disegno di politica economica in Europa. In Europa i Governi sono convinti che il futuro del nostro continente non può essere un futuro di crescita fintanto che non si consolida la stabilità finanziaria. Il documento indica un vincolo preciso: la stabilità finanziaria è l'elemento dominante su cui aggregare la volontà di tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea.

finanziaria è l'elemento principale, il cardine su cui costruire le nostre scelte di politica economica e finanziaria per il futuro? Badate bene, la stabilità finanziaria (e qui entra in gioco una riflessione sulla storia del nostro Paese e sull'attualità del nostro Paese), come dice il documento, è una entità complessa e, diversamente da come si sosteneva nella fase pre-crisi, quando all'ordine del giorno c'era

per la prima volta - ritengo anche e soprattutto per iniziativa del Governo italiano - la stabilità finanziaria va considerata non solo avendo riguardo agli equilibri di finanza pubblica, ma anche alla sostenibilità della finanza privata, agli equilibri di finanza privata, e nel documento - lo dico ai colleghi talvolta distratti - si fa esplicito riferimento al risparmio accumulato dalle famiglie,

nella crisi, fino ad oggi, ha retto meglio di altri Paesi, perché è un Paese diverso degli altri. Da noi le famiglie, negli anni, hanno saputo accumulare risparmio la presenza delle piccole e medie imprese è un *asset* fondamentale in queste condizioni; la tenuta, la solidità e la patrimonializzazione del sistema bancario è un fatto unico che rende questo sistema il più forte in Europa. Però tutte queste cose

che considerare la stabilità finanziaria in questo modo, nei fatti, ci premia perché ci mette in una condizione migliore rispetto a tanti altri Paesi. Se conveniamo allora su questo dovremmo convenire, perché è una scelta condivisa a livello europeo, sui processi che l'Unione europea ha indicato: la riforma globale del sistema finanziario (che riguarda più gli altri Paesi che l'Italia, perché l'Italia l'ha fatta alla fine degli anni Ottanta); la sorveglianza fiscale con la revisione del Patto di stabilità e crescita (occorre inventare nuovi strumenti per garantirci nella crescita) e la sorveglianza macroeconomica per superare le criticità economiche di ogni sistema produttivo e quindi anche del nostro. Se le premesse le premesse sono queste, e se si conviene sulle stesse, dovremmo, subito dopo, convenire anche sul fatto che questa disputa tra i difensori rigoristi della stabilità finanziaria e coloro che affermano che ci vuole la crescita non esiste,

averlo fatto, possiamo pensare a mettere in campo quelle decisioni di politica economica che favoriscano la crescita attraverso il recupero della competitività di un sistema che necessita di essere riformato. Quindi, non più una crescita collegata al ricorso a deficit pubblici, ma un chiaro messaggio all'esterno di questo Paese per dire che non potremo mai più contare in futuro su risorse pubbliche in eccesso, perché il bilancio statale sarà quello che sarà, perché il debito pubblico lo abbiamo e perché questo vincolo è un dato irremovibile e fondamentale che dobbiamo tener presente.

della crescita lo dobbiamo tenere ben presente. Su questo noi della Commissione infrastrutture abbiamo anche questa mattina riflettuto, come lo abbiamo fatto nelle settimane scorse, e diciamo che certamente le riforme che non costano vanno fatte e vanno realizzate in sintonia

mi sembra un documento aperto, proprio perché, come è stato detto all'inizio, è una bozza, ritengo di dover portare un contributo che è anche quello della Commissione che ho l'onore di presiedere. Assieme al vincolo irrinunciabile, assieme agli obiettivi (la questione meridionale, la questione fiscale, la questione nucleare e la questione legale) certamente, per recuperare competitività, non possiamo ignorare la questione infrastrutturale.

Mettere in condizione i privati di fare ciò che possono fare nell'attuale condizione del nostro sistema produttivo vuol dire credere nei nuovi strumenti che abbiamo approntato, credere nel *project financing* di terza generazione ed immaginare, attraverso un salto culturale che tutti insieme dobbiamo compiere, compiere, che tutte le infrastrutture che hanno una capacità di reddito devono essere progettate, costruite e gestite dagli operatori privati che solo attraverso la gestione possono recuperare

concordemente, anche se è difficile far ciò in un Paese che negli anni passati ha chiesto sempre tutto al bilancio dello Stato, che ha sempre immaginato che i più bravi fossero quelli che riuscivano ad attingere più degli altri negli apparati dello Stato, nella centralità dei Ministeri

Dobbiamo avere il coraggio, laddove non esistono risorse pubbliche, di agire sulla tariffa. Il populismo non paga nell'Europa del rigore. la capacità ed il coraggio di compiere alcune scelte coerenti e coraggiose che credo possa fare, meglio di altri, un Governo con una maggioranza di centrodestra.

Un paragrafo breve e quasi nascosto verso la fine del documento. E con buona ragione, direi, perché i dati, naturalmente non citati nel testo ma solo nella tabella sottostante, sono terribili: ben il 18,7 per cento degli italiani è a rischio di povertà! Nel testo tuttavia, a mo' di consolazione, si dice che: «la situazione italiana non si discosta molto dalla media europea». Subito dopo aver letto (nelle note e non nel testo) che «È la difficoltà di trovare un'occupazione che spiega i livelli di povertà elevati: è povero il 26,7% (...) delle famiglie con a capo una persona in cerca di lavoro» si apprende che il Governo intende perseguire l'impegno di riduzione dell'area della povertà «sia attraverso trasferimenti monetari o equipollenti (...), sia intervenendo con politiche attive che promuovano l'elevazione dei tassi di occupazione». per quanto riguarda i «trasferimenti monetari o equipollenti», mi sembra sufficientemente significativo il fatto che l'unico esempio citato sia la *social* *card*, cioè uno strumento che tutte le indagini più serie hanno dimostrato essere stato un clamoroso fallimento. Vi sono poi le politiche attive che promuovono l'elevazione dei tassi di occupazione» che, si suppone, dovrebbero essere quelle citate nel paragrafo precedente. Un testo davvero sorprendente, un vero libro dei sogni che descrive politiche mai attuate, oppure che sono foriere di gravi effetti sul mondo del lavoro ma che vengono portate avanti solamente per motivi di pura ideologia. Fra le azioni riformatrici vengono infatti citati il collegato lavoro, il piano triennale adottato a luglio, la formazione. Sul collegato lavoro ci siamo ampiamente dilungati durante le numerose ed estenuanti letture parlamentari che ne hanno caratterizzato l'*iter.* Qui è sufficiente ribadire che quell'accozzaglia di norme incoerenti e giustapposte è ben lontana dal potersi definire «azione riformatrice» e il massimo vantaggio che potrebbe portare al sistema è di non produrre che pochi e limitati effetti pratici. Quanto alle ormai famose disposizioni sulla conciliazione e l'arbitrato, com'è stato detto da tutta la più autorevole dottrina, non faranno altro che far aumentare il contenzioso, sempre che non vengano spazzate via prima per la loro incostituzionalità. Il piano triennale per il lavoro individua tre priorità: lotta al lavoro irregolare e aumento della sicurezza sul lavoro, decentramento della regolamentazione, sviluppo delle competenze per l'occupabilità. Quanto alla prima, forse si sarebbe dovuto più brevemente e correttamente scrivere «lotta alla sicurezza sul lavoro», visto che dall'inizio della legislatura il Governo è applicato con costanza nello smantellamento delle tutele previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, da ultimo con il cosiddetto disegno di legge sulla semplificazione. Il massimo sforzo è stato la realizzazione di una costosa e falsa campagna propagandistica, dove con lo slogan «Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene» si è cercato di scaricare la responsabilità della prevenzione degli infortuni e delle cosiddette morti bianche sui soli lavoratori. Il decentramento della regolamentazione si è tradotto nella distruzione delle garanzie contrattuali, nella ricerca sistematica della divisione delle forze sociali e nella promozione degli accordi separati, nel ritorno alla diffusione della precarizzazione, con il risultato che oggi milioni di lavoratori, soprattutto giovani, si trovano con un presente incerto e privi di qualunque prospettiva per il futuro. Quanto allo sviluppo delle competenze per l'occupabilità, che prevedrebbero la valorizzazione dell'azienda come luogo di formazione, forse è in tal senso che vanno lette norme assurde, come quella contenuta all'articolo 48 del collegato lavoro, che dietro il paravento della formazione nascondono l'abbassamento surrettizio dell'età scolare. Del resto, dal 2008 ad oggi, riguardo ai trasferimenti di risorse da destinarsi al settore dell'istruzione, tutte le leggi finanziarie fin qui approvate - ultima la legge di stabilità in corso di approvazione - hanno previsto e prevedono significativi tagli. La finanziaria 2009, oltre che confermare tutti i macroscopici tagli introdotti dal decreto-legge n. 112 del 2008, ha anche provveduto a ridurre il fondo per l'offerta formativa di ben 29 milioni, portandolo a soli 150, contro i 274 della sua consistenza originaria, prevista per sostenere anche la formazione del personale, l'assistenza ai portatori di handicap, l'innovazione e l'alternanza scuola-lavoro. Progressivamente il fondo in questione è stato ulteriormente ridotto a 130 milioni nel 2010 ed è prevista una dotazione di soli 99,5 milioni, sia per il 2011 che per il 2012. Nella sezione 3.2 del Programma nazionale di riforma si citano «le riforme attuate - quella scolastica - e quelle in corso di attuazione - quella universitaria», nonostante non sia stata ancora introdotta nell'ordinamento alcuna legge di riforma risulta essere ad oggi il famigerato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008: un intervento volto esclusivamente al contenimento delle spese, nonché censurato dal Consiglio di Stato, in quanto non rappresenta altro che un decreto-legge di natura esclusivamente economica, volto a deprimere ulteriormente il già precario sistema formativo italiano, mentre il Governo continua a chiamarlo riforma della scuola. Anche il decreto-legge n. 137 del 2008, lungi dal rappresentare una riforma del settore dell'istruzione, ha introdotto poche e discutibili norme riguardanti l'istruzione primaria, fra le quali ricordo la reintroduzione del maestro unico, la cui applicazione fatti disattesa perché non rispondente alla richiesta delle famiglie Quanto alla riforma dell'università, il cui obiettivo primario è indicato nell'eliminare «la frammentazione degli indirizzi» al fine di usare più efficacemente le risorse, ad oggi risulta approvato dal Parlamento il solo decreto-legge n. 180 del 2008. Sappiamo che il solo Senato si è pronunciato fino ad oggi e attualmente questa riforma è ferma alla Camera per assenza di copertura finanziaria. Ed è proprio questa la drammatica realtà. Come ha detto con efficace sintesi il ministro Galan, non c'è una lira. Del resto, dopo due anni di nessuna scelta o di scelte sbagliate, francamente non c'era da aspettarsi qualcosa di diverso. La sola consolazione per noi è che chi ha provocato tutto ciò sembra finalmente essere arrivato al suo capolinea politico. *(Applausi

l'Europa degli ultimi anni è sfidata sia nella produzione della ricchezza che nel suo modello sociale. Grandi Paesi di antiche civiltà hanno impresso a loro stessi ritmi di crescita molto più elevati di quelli europei e hanno con ciò cambiato profondamente non solo i loro rapporti con l'Occidente e con l'Europa, ma li hanno altresì sollecitati a ridefinire sé stessi. L'Europa, dopo un primo periodo di smarrimento, in cui i Paesi hanno spesso pensato di potercela fare meglio da soli, cerca ora una nuova definizione di sé attraverso un progetto comune in grado di rilanciare la produzione di ricchezza e il proprio modello sociale. L'Europa ci dice: possiamo farcela se compiamo una svolta. Nei decenni passati l'Europa ha potuto costruire se stessa e spazi comuni prescindendo molto da ciò che avveniva fuori dai suoi confini, in Asia, in America Latina e nella stessa Africa. Oggi questo non è più possibile o meglio non è più possibile se l'Europa vuole essere un continente forte e competitivo per ciò che produce, per come lo produce e per i risultati che ottiene. I ripiegamenti nazionalisti, territoriali, comprensibili come prima reazione all'avanzare della forza degli altri Paesi, oggi sarebbero suicidi se i territori e i Paesi non sono ricompresi e ridislocati in politiche di sistema. L'Europa può accettare la sfida se nella globalizzazione rispetto a Paesi di miliardi di esseri umani in crescita si presenta unita, con un progetto forte e un modello sociale altrettanto forte. La sfida europea ha bisogno di Paesi europei forti. Per l'Italia la sfida è doppia perché il suo sistema, crescita, pubblica amministrazione, innovazione, *welfare* inclusivo, è in forte affanno e presenta dei vistosissimi segni di declino. L'Italia è il penultimo Paese al mondo per crescita economica, l'ultimo per tasso demografico. Da questi due dati occorre partire. Una visione economicistica non salva il nostro Paese dal declino. Una riduzione del debito, indispensabile per la stessa equità sociale, se non si avvale di politiche espansive non muoverà quelle risorse umane in grado di fare la differenza in termini di crescita. in riferimento a ciò, occorre dire che la maggioranza non ha presentato una bozza convincente, adeguata per attrezzare l'Italia alla sfida europea. La nostra crescita non potrà avvenire

L'onorevole Prestigiacomo ieri parlava di «*welfare* dei nonni». Non è un riconoscimento di importanti figure parentali, ma l'opposto. È gettare anche sui nonni, mentre si taglia il fondo per la non autosufficienza, l'incapacità di promuovere un *welfare* per lo sviluppo del Paese. Cosa ha impedito ed impedisce all'Italia di investire sulle donne e sulle nuove generazioni? Lo impedisce una visione arretrata e ripiegata su se stessa. Dice Ferrera in un recente articolo: «L'incremento dell'occupazione femminile nei Paesi sviluppati ha contribuito alla crescita globale più dell'economia cinese. Peccato che l'Italia non abbia fatto nulla per inserirsi in questo circuito positivo. E dire che sarebbe bastato investire 2 miliardi di euro in una rete di asili nido per avere ricadute positive». Ecco, l'Italia non solo non fa questo, ma anzi da questa finanziaria si tolgono 100 milioni di euro per il piano straordinario sui nidi

questo modo l'intera spesa sociale in pochissimi anni è stata drasticamente ridimensionata. Soltanto nel 2011, rispetto al 2010, si determina Eppure anche in Italia le esperienze regionali hanno mostrato la stretta connessione tra servizi all'infanzia e occupazione femminile. La riforma dei servizi all'infanzia ha un grande valore. Si può fare, abbiamo una legge d'iniziativa popolare che ha raccolto oltre 200.000 firme, e a cui hanno dato un contributo le migliori forze del Paese. Sull'investimento, non solo finanziario, sull'infanzia e sull'adolescenza è in atto una grande regressione culturale. Di più, si comincia a smarrire l'importanza della tutela e della promozione della persona in via di sviluppo. È in atto una precocizzazione, una "adultizzazione", tutta a beneficio di una mancanza di responsabilità verso le tappe della crescita. Da un lato, vi è il clamore e le adolescenti vengono messi al centro e, dall'altro, vi sono voyeurismo e consumismo della giovane età, non protezione, non promozione, non rispetto e spesso consumo. Questo è il significato dell'adultizzazione. La richiesta della precocizzazione è frutto di un narcisismo di classi dirigenti non responsabili verso le nuove generazioni. Secondo i dati OCSE noi spendiamo lo 0,65 per cento per l'infanzia e l'adolescenza (la Francia, ad esempio, ne spende tre volte tanto), con grandi diseguaglianze tra Nord e Sud. Sud. La questione principale è investire per i nidi, per la povertà minorile, contro la dispersione scolastica. Abbiamo votato contro il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ma la stessa maggioranza ha espresso critiche rilevanti

che la maggiore inclinazione alla depressione nasce dal contrasto tra la loro aspettativa di crescita e di sviluppo e il venire meno di quelle del contesto in cui vivono e del Paese. Ecco, un forte Paese dovrebbe partire da questo. Se già da giovanissimi le ragazze e i ragazzi italiani non hanno fiducia nel loro futuro, allora anche l'Italia non potrà affrontare nessuna sfida importante. Se vogliamo ricominciare a crescere, scommettiamo anche sulla loro fiducia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

I termini del nuovo Patto di stabilità, sebbene non ancora definiti nei dettagli, possono comportare diversi scenari di evoluzione della nostra economia nei prossimi decenni, ma tutti questi scenari si prefigurano come «lacrime e sangue». Quando un debito pubblico, come quello italiano, raggiunge le dimensioni attuali del 108,5 per non è probabile che un programma vincolante di ordinato rientro entro il 60 per cento del PIL possa realizzarsi in 20 anni senza un progressivo impoverimento del Paese. Per sfuggire a questa dura realtà occorrerebbero eventi straordinari, come un balzo in avanti nella crescita, o una fiammata di inflazione, o un'operazione di finanza straordinaria, o tassi di interesse permanentemente su valori minimi, che sono tutti eventi irrealizzabili irrealizzabili nell'attuale assetto della nostra integrazione nell'Unione economica e monetaria. L'alternativa a disposizione sul piano interno dovrebbe essere un radicale rinnovamento dell'economia che la ponesse in grado di correre, invece di trascinarsi come avvenuto negli ultimi 15 anni; ma quanto sia fattibile è un interrogativo senza risposta. Quale che sia la definizione finale del nuovo Patto di stabilità - i cui elementi quantitativi non sono ancora noti

una conclusione è chiara: qualsiasi riduzione sostenibile del debito pubblico italiano è possibile solo comprimendo la spesa primaria e operando per un rapido ritorno ad una crescita elevata e duratura. Quali sono le due vie di fuga? La prima è ottenere dall'Unione europea uno stretto coordinamento delle politiche economiche che obblighi i Paesi in *surplus* di bilancia corrente con l'estero, segnatamente la Germania, a perseguire politiche di riflazione della domanda interna.

che questo documento sia solo l'avvio di un dibattito e di confronto, altrimenti avrebbero ragione autorevoli esponenti dell'opposizione nel dire che si è trattato di una sommatoria raffazzonata dai Ministeri, di contributi, perché questa è l'unica via di uscita che abbiamo all'interno per tentare di riportare il Paese ad una crescita economica. Tuttavia, visto il fallimento dell'Agenda di Lisbona, dobbiamo chiederci - e dovrebbe chiederselo il Ministro dell'economia e delle finanze - quali sono le riforme strutturali che non hanno costo e perché in un documento come questo non compare un elenco di riforme senza costo. Esistono riforme senza costo? Questa è una domanda preliminare, perché se non esistono riforme senza costo

perché quei vincoli sono pesanti, che neppure il Governo credo conosca, né quest'Aula. Sono vincoli quantitativi ignoti a tutti,

lanciare grida di dolore sugli investimenti in questo o quel settore. Il problema è stabilire un rapporto tra i vincoli di bilancio e quello che è possibile fare se ci sono riforme *no cost*. Quelle devono e possono avere una precedenza assoluta. Se questo metodo non sarà possibile allora il nostro Paese è condannato ad una inesorabile decadenza. Questo lo dico con amarezza perché condivido il grido di dolore del senatore Morando sulla fretta, sul pressappochismo di alcuni documenti

che la responsabilità è oltre che della classe dirigente anche del mondo dell'informazione. Ieri quelle tribune erano affollate. Oggi non c'è nessuno. *(Applausi dal E allora, senatore Morando, se è vero quanto lei ci ha detto, cioè che il cancelliere Merkel ha risposto per sette ore - ed è vero - e se è vero che all'Assemblea nazionale francese

al Programma nazionale di riforma, significa che la decadenza non riguarda soltanto la classe politica e che c'è una colpa anche del mondo dell'informazione.

un fondo di comune analisi ed anche, in obiettivo finale, la comune soluzione dell'obiettivo. Questo è trasparso anche dalla pregevole relazione del relatore di minoranza Morando. Morando. Certamente, il percorso è diviso anche dall'appartenenza. È vero che il ruolo dell'opposizione è quello di dire che il Governo fa ed ha fatto poco, e ci sarebbe da stupirsi se fosse altrimenti, ma non dobbiamo cadere nello sport nazionale di denigrare il nostro Paese ad ogni occasione. Non è però comunque denigrare il constatare le realtà. Molto è stato fatto e non lo ripeterò (pensioni, federalismo, servizi pubblici, semplificazione, scelta nucleare, piano della logistica, piuttosto che università e lavoro), molto, certamente, rimane da fare. Credo, colleghi, che proprio nell'ottica della competitività internazionale uno sforzo lo dobbiamo e lo possiamo fare tutti, a cominciare dal fatto di discutere di merito nei vari provvedimenti e non solo di salvaguardie, e molti interventi hanno La riforma dell'università è per avere laureati più preparati, per avere una scuola che funzioni, non per salvare qualche professore o ricercatore. se discutiamo di giustizia non è per garantire carriere, né procedure che diano lavoro agli appartenenti all'ordine forense, ma è per dare giustizia ai cittadini. Certo, lo hanno affermato diversi colleghi: non vi sono fondi per interventi pubblici rilevanti, anzi è necessario ridurre le spese per portarci almeno in avanzo primario e, con ciò, non aumentare l'ingente debito pubblico ha. Tuttavia, credo che il Programma nazionale di riforma presentato dal Governo, tenendo ben presente questo vincolo, dia percorsi, indirizzi e spazi per un'azione che può portare il nostro Paese a superare le difficoltà esposte e riprendere la via dello sviluppo. È possibile sviluppare una politica di mercato, di merito e di competizione anche senza intaccare le garanzie sociali per le situazioni più deboli. sono in contrasto libero mercato e Stato sociale, sono in contrasto libero mercato e assistenzialismo: quando le nostre PMI e in particolare i piccoli imprenditori devono pagare imposte, tasse e contributi, sommando quindi tutta questa fiscalità, che va oltre il 60 per cento del proprio credito, sono demotivati a fare; ma è anche demotivato l'imprenditore che vede l'assenteismo ad un tasso percentuale doppio dell'Europa e un dipendente pubblico non licenziabile anche se lavativo. Non si intaccano diritti civili, ma diritti di parassitismo che si sono creati nel tempo. Colleghi, credo che la maggioranza degli italiani - e non mi riferisco a quelli che votano a destra o a sinistra, al Sud o al Nord si renda conto delle difficoltà, possa accettare sacrifici, ma non possa andare oltre nell'accettare la difesa ad oltranza di parassitismo e burocrazia. Si è parlato dei vincoli, di rigore e di riforma. Una notazione anche per i più disattenti o gli assenti durante la discussione: sovente in quest'Aula si discute della copertura di norme per pochi milioni di euro;

Vorrei ricordare ai colleghi che l'1 per cento di quel miliardo di euro giornaliero che collochiamo è

è fondamentale fare le riforme e, in questo caso, esse devono avere una valenza di costo minore ed effetti maggiori per lo sviluppo. Per questo motivo, signor Presidente, colleghi, io il Programma nazionale di riforma dia i giusti indirizzi di azione coordinata, che saranno discussi nell'ambito dell'Unione europea, per lo sviluppo del nostro Paese.

metodologia con la quale stiamo seguendo la fase di preparazione della bozza di Programma nazionale di riforma e sui tempi della nostra discussione. Sono osservazioni fondate; tuttavia, alcuni dei senatori intervenuti a questo proposito hanno argomentato le loro valutazioni critiche sulla ristrettezza dei tempi sulla base di una valutazione che, invece, io radicalmente non condivido. È la valutazione relativa al fatto che non esisterebbe, per il Governo italiano, come per gli altri Governi europei, nessun vincolo giuridico alla presentazione della bozza di Programma nazionale di riforma il 12 novembre prossimo.

*spread*, del differenziale dei titoli di Stato tedeschi rispetto a quelli italiani nel corso di queste giornate di sostanziale apertura della crisi di Governo. L'andamento è assai preoccupante; e voi immaginate cosa accadrebbe se il Governo italiano non presentasse il 12 novembre,

il 12 novembre, possibilmente al mattino presto, la bozza di Programma nazionale di riforma. Se poi dovessi scriverla io, la scriverei diversamente da come l'ha scritta il Governo, e questo lo si vedrà sulla base delle valutazioni

a causa del modo con cui il Governo si sta rapportando al Parlamento e - fatemi aggiungere, colleghi - al Paese su questa fase di rielaborazione della *governance* economica europea, compresa l'elaborazione della bozza del Programma nazionale di riforma, quale forza politica trae il Governo italiano nel confronto con gli altri Governi a livello europeo, nelle sedi comunitarie, da questo tipo di coinvolgimento, che implicitamente emerge dalle valutazioni critiche che molti di noi hanno fatto a proposito della metodologia della nostra discussione? È chiaro: il Governo sta rinunciando, con questo sequestro delle informazioni e con questa sottovalutazione della portata straordinaria delle innovazioni che sono di fronte a noi nella costruzione di una nuova *governance* europea, europea, a trarre da un positivo rapporto con il Parlamento ed il Paese la forza necessaria per fare prevalere nella definizione delle nuove scelte di politica di bilancio e di politica economica in Europa diciamolo con chiarezza - gli interessi nazionali compatibili con il quadro di riferimento europeo. È una valutazione che merita molta più attenzione di quanto mediamente le stiamo dedicando, perché perché la forza dei Governi europei, anche nel confronto europeo, deriva dalla loro capacità, quando esprimono una posizione, di rendere chiaro all'interlocutore che quella posizione è posizione è maturata con un rapporto positivo con il loro Paese e con i portatori di interessi economici e sociali. Tutto questo manca all'Italia, a causa della crisi politica del Governo di centrodestra e a causa del fatto che il principale protagonista di questo confronto, cioè il Ministro dell'economia, elude ed evade rispetto al confronto con il Parlamento e il Paese sulle scelte che dobbiamo compiere. secondo luogo, il senatore Grillo e molti altri hanno sottolineato la preoccupazione che riguarda il rapporto che deve sempre essere mantenuto tra tra le politiche di consolidamento del debito pubblico, le politiche di rigore - come le chiamiamo nel nostro dibattito interno di politica economica - e le politiche per la crescita. Se ho capito bene, egli ha manifestato preoccupazione che da parte nostra ci sia un'incertezza su questo punto. Evidentemente, non ha ascoltato né la relazione né molti degli interventi che abbiamo fatto, perché esattamente sulla definizione del sentiero sottilissimo che sta tra politiche di consolidamento della finanza pubblica e politiche per la crescita abbiamo sviluppato la nostra proposta. Quindi, senatore Grillo, tutta la maggioranza e il Governo devono essere tranquilli: per quello che riguarda l'opposizione del Partito Democratico, noi non stiamo proponendo affatto - basta leggere la proposta di risoluzione - politiche di sfondamento dei conti. critichiamo il Governo per non avere ancora con la necessaria determinazione definito un piano rigoroso di ricostruzione dell'avanzo primario, in maniera da rendere credibili gli obiettivi, molto ambiziosi, di riduzione progressiva del volume globale del debito pubblico, in un contesto di riforme che rilancino la produttività del

dei mercati e dei fattori fondamentali di produzione, dal lavoro fino ai servizi, alle libere professioni, Si tratta di riforme che non costano, ma sono essenziali per elevare la produttività totale dei fattori perché riformano profondamente i mercati fondamentali dei fattori. Proprio per questo, la mia domanda è: Governo, maggioranza, relatore della maggioranza, che rapporto di coerenza c'è tra quello che avete scritto nel documento, pur molto insufficiente, a proposito di riforma del mercato delle professioni liberali per aumentare la capacità competitiva del Paese, e il disegno di legge che tra qualche minuto riprenderemo a discutere sulla riforma della professione forense? Sono due ipotesi che vanno in una linea completamente alternativa tra di loro. C'è una riforma della professione forense ispirata ad obiettivi di chiusura e di ribadimento di questo settore dentro un contesto che è quello corrispondente - e allora funzionava - all'economia agricola. Sono stati i dottori commercialisti, non esattamente noti come grandi liberalizzatori (com'è noto), a redigere un documento in cui hanno sottolineato che stiamo riorganizzando o pretendiamo di riorganizzare il mercato delle professioni liberali ragionando come se l'economia italiana, dentro cui ospitare questa riforma, fosse l'economia agricola di cento anni fa. fa. Vi volete decidere a mettere in mora il disegno di legge sulla professione forense, per renderlo coerente - perché di riforma c'è bisogno - con il disegno di riforma dei mercati fondamentali e dei fattori che dobbiamo presentare in Europa? Se continuate così, la credibilità vostra e del Paese nel suo complesso in Europa finisce sotto le scarpe, per una ragione molto elementare: nel programma scrivete una cosa

nella strategia generale per l'occupazione c'è una scelta chiave da fare (una volta tanto, nel documento, c'è la sottolineatura di una priorità, cosa che non accade quasi mai). Qui c'è: si dice che la priorità è l'incremento del tasso di occupazione femminile. Io sono molto d'accordo con questa sottolineatura, perché, nel contesto di una politica che voglia utilizzare le principali risorse oggi inutilizzate per una strategia di rilancio dello sviluppo, è abbastanza evidente che la fondamentale e la principale delle risorse oggi inutilizzate consiste nella volontà, nella capacità di lavoro, nella voglia di fare e nell'intelligenza di milioni di donne che vorrebbero lavorare anche fuori casa, ma non ci riescono, a causa della chiusura della realtà economica del Paese, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Studiano meglio dei ragazzi coetanei, ottengono migliori risultati, si impegnano di più, sono più responsabili, ma noi rispondiamo con un tasso di occupazione e di partecipazione delle donne alla forza lavoro da Paese del terzo mondo. Questo è il dato, ed è giusto sottolineare la priorità. Ma vi volete decidere, una volta sottolineata questa priorità, che condividiamo tutti, ad indicare quali sono le scelte fondamentali che immediatamente riequilibrano le opportunità di lavoro a favore delle donne e a danno dei maschi? È chiaro che qui non c'è il Bengodi: continuiamo a fare come abbiamo fatto oggi, e le donne aumenteranno nel loro numero di partecipazione alla forza lavoro non si sa quando. Allora, due cose precise: in primo luogo, il credito di imposta automatico per le nuove assunzioni di donne nel Mezzogiorno. Non è vero che la Commissione europea lo impedisce:

In secondo luogo, noi abbiamo presentato un disegno di legge che - sissignori - riduce le aliquote IRPEF del reddito da lavoro delle donne, a parità con quello di un maschio, allo scopo di riequilibrare, attraverso questa misura, le minori e peggiori opportunità che hanno le donne sul mercato del lavoro rispetto ai maschi. Vogliamo compiere nel Programma nazionale di riforma una scelta strategica di questa portata, orientata a favore della componente fondamentale che può essere utilizzata tra le risorse del Paese per la promozione per la promozione dello sviluppo? Nel Programma nazionale di riforma si cita l'esigenza, ma non si fornisce alcuna risposta, il contrario di quello che un Programma nazionale di riforma serio dovrebbe fare. Vedete, colleghi, anche il colleghi, anche il vostro documento, per carente che sia, conferma un punto che io considero assolutamente cruciale e che dovrebbe essere la base per il rapporto tra la politica e il Paese in una chiave, sissignori, pedagogica, perché la politica ha una funzione pedagogica e di guida rispetto al Paese se vuole essere politica, quella con la "P" maiuscola che in Italia abbiamo da tempo smarrito. *(Applausi abbiamo la prova che le riforme strutturali pagano. Il senatore Grillo ha giustamente citato tra i fattori di forza, che vengono citati anche nel Programma, il nostro il nostro sistema bancario. Ma perché il nostro sistema bancario è relativamente forte a paragone con quello degli altri Paesi europei? Nel 1992 e poi negli

Si dice che abbiamo una spesa pensionistica per il futuro più in equilibrio di altri Paesi europei, ed è vero. è vero. Siamo in questa situazione assolutamente positiva. Ma perché ci siamo? Perché nel 1992 il Governo Amato, nel 1995 il Governo Dini, nel 1996 il Governo Prodi e - diciamolo chiaramente - nel 2010, il Governo Berlusconi hanno fatto riforme strutturali che hanno messo sotto controllo la spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo. Le riforme pagano. E questa è la base da cui partire al Paese quelle riforme che nell'immediato producono problemi, come hanno prodotto problemi la riforma previdenziale e quella del sistema bancario, ma attrezzano il Paese ad essere pronto

Innanzitutto, come giustamente è stato detto, questo piano di riforme va nell'ambito di un nuovo quadro europeo di indirizzo comune e di politica economica che deve portare all'obiettivo prioritario, quello della riduzione del debito. In Europa, come si è discusso la settimana in questa Aula, siamo riusciti ad introdurre altri parametri di valutazione delle *performance* di un Paese; ricordiamoci però che la riduzione del debito pubblico è l'obiettivo prioritario prioritario di tutti i Governi europei per la salvaguardia finanziaria degli Stati membri dell'Europa e della moneta unica. Nell'ambito di questo quadro, il piano delle riforme deve fare quello che il senatore Morando ha citato come una maratona su un filo d'acciaio, che è un'espressione che sposa benissimo l'azione che deve essere fatta che deve essere fatta cercando di esaltare i punti di forza del nostro Paese, di ridurre i punti di debolezza, e di far tutto questo non utilizzando l'incremento della spesa pubblica come benzina per poter attuare questo obiettivo. Quindi, tutto deve essere fatto a costo zero, innanzitutto cercando di riqualificare la spesa: il primo grande obiettivo che abbiamo, infatti, è proprio questo, per cercare di far sì che si utilizzi

maggiore utilizzo dei fattori produttivi che possono cercare di fornire uno stimolo. Nello stesso tempo, riteniamo che su alcuni settori si debba assolutamente fare chiarezza e, quindi, ci si debba orientare

un fattore produttivo più utile alle imprese che competono sul mercato mondiale, bisogna fare, ad esempio, scelte come quella sul nucleare. Chiediamo pertanto che anche

merito a tutti i settori e che quando si parla di scuola e università, elementi fondamentali per lo sviluppo del nostro futuro, si pensi veramente

*(FLI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'introduzione del semestre europeo è uno degli aspetti forse più innovativi della riforma della *governance* economica nell'area dell'euro. Esso comporta cambiamenti incisivi in tema di programmazione economica e finanziaria anche in Italia. Questi cambiamenti riguardano sia la tempistica dei documenti programmatori e delle decisioni, sia i contenuti dei documenti stessi. Sotto quest'ultimo profilo, uno dei risvolti più importanti e senza dubbio più positivi di questa riforma è proprio quello di avere conferito al Programma nazionale di riforma il giusto peso nell'ambito del ciclo di programmazione della politica economica. Nel nuovo assetto di programmazione al PNR viene riconosciuto il rango di altri documenti di programmazione, come la Decisione di finanza pubblica, approvata dal Parlamento giusto un mese fa e che sostituisce il tradizionale DPEF, e il Programma di stabilità, i quali sono stati da sempre il punto quasi esclusivo di riferimento per la valutazione della nostra strategia di politica economica in sede europea. La vecchia Strategia di politica economica europea era però basata sulla sola gamba del rigore finanziario, che ha consentito all'Italia, come ad altri Paesi, di conquistare una sostanziale stabilità dei conti pubblici e la credibilità nei confronti dei mercati finanziari, ma che ha tuttavia mostrato i propri limiti.

È quindi maturata la consapevolezza che non basta avere azioni mirate esclusivamente alla stabilità delle finanze pubbliche; occorre avere una struttura più forte per il coordinamento di tutte le politiche economiche di riforma, che devono rispondere ai reali bisogni dei Paesi, affrontare con efficacia gli ostacoli allo sviluppo eliminando i nodi strutturali e i colli di bottiglia. È questa consapevolezza che ha dettato la scelta del Consiglio europeo di adottare la nuova Strategia «Europa 2020». Con il PNR, perciò, anche quelle politiche economiche strutturali, fondamentali per il rilancio del sistema Paese e della crescita economica, ora acquistano finalmente il proprio spazio di discussione in fase di programmazione economica e finanziaria. Il PNR diventa un tassello fondamentale nella strategia di politica economica del Governo, ma anche un banco di prova su cui l'Italia misura la propria credibilità in sede europea. Questo documento rappresenta la mappa che il Paese dovrà seguire per raggiungere obiettivi di crescita e occupazione, che, a nostro avviso, sono ineludibili, e in questo senso noi lo vogliamo considerare anche un primo, importante segnale a testimonianza della volontà di rilancio del Governo, dopo una lunga fase di stallo e di incertezza sul piano dell'economia. In un momento in cui, non solo al Governo, ma all'intera classe politica viene chiesto a gran voce di tornare ad occuparsi di ciò che veramente conta per il Paese, il PNR rappresenta una occasione di dialogo tra Governo e Parlamento da non sprecare, al fine di individuare i problemi dell'Italia e le azioni necessarie a risolverli. Sul PNR l'Esecutivo può e deve tornare a confrontarsi con il Paese per il bene dei cittadini e la competitività delle imprese. È una sfida da accettare e vincere. *(Brusìo).* Signor Presidente, vorrei ricordare che chi non ha interesse al dibattito può uscire: non c'è un obbligo all'ascolto. Nel merito, condividiamo la filosofia e la logica di fondo espressa nel documento di perseguire la crescita economica senza far ricorso a nuova spesa pubblica corrente, ma facendo leva esclusivamente sugli investimenti e sulle riforme strutturali, le sole capaci di migliorare la competitività del sistema Paese. È essenziale concentrare gli sforzi e le risorse disponibili,

e questo è ancora più vero nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. In secondo luogo, il fisco, perché il Paese ha bisogno di riformare il proprio sistema fiscale, anche qui non solo perché occorre ridare respiro all'economia riducendo l'enorme carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, ma anche perché riformando il fisco si fa il passo più importante nel ridisegno dei rapporti tra Stato e cittadini. In terzo luogo, l'energia, affermando ancora una volta che la scelta del nucleare è cruciale per l'Italia, perché assicura il soddisfacimento del fabbisogno energetico di un Paese che vuole tornare a crescere e garantire benessere e sicurezza a tutti i propri cittadini. Infine, l'assetto normativo-istituzionale, perché è l'*humus* sul quale crescono i rapporti economici e sociali di un Paese sviluppato, civile e democratico. Gli obiettivi fissati per il 2020 sono talmente ambiziosi da richiedere un deciso cambio di marcia in tutti i settori. Per questo, pur condividendo l'impostazione generale del documento e il significato potenziale che esso ha in termini di rinnovato impegno del Governo, vogliamo richiamare l'attenzione su altri temi importanti sui quali sarebbe opportuno che la versione definitiva del Programma presentato alla Commissione europea si soffermasse in modo più incisivo, delineando con maggiore chiarezza le prospettive e le azioni di politica economica proposte dal Governo. Anzitutto, le politiche per la ricerca e l'innovazione, che devono tener conto della struttura produttiva del Paese composta in prevalenza da piccole e medie imprese le quali, senza un adeguato sostegno del sistema pubblico di ricerca in particolare sotto il profilo dei trasferimento tecnologico, non possono fare innovazione e quindi competere alla pari sui mercati globali. Proprio per questo è essenziale attivare un grande piano sinergico di investimenti nella costruzione di un sistema a rete che coinvolga in modo efficace ed efficiente scuola, università centri di ricerca e mondo delle imprese. Sempre in tema di innovazione tecnologica non dimentichiamo poi la fondamentale importanza di garantire, nell'epoca in cui i rapporti economici e sociali sono dettati dall'informazione e dalla comunicazione digitale, tutti abbiano la concreta possibilità di accedere a Internet. Per questo il progetto di portare la banda larga finalmente in tutto il Paese è un obiettivo irrinunciabile, anche perché dobbiamo adeguarci agli obiettivi fissati a livello comunitario dall'Agenda digitale europea. Una politica per il rilancio della ricerca e dell'innovazione è fondamentale anche per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno dove la creazione di centri di eccellenza può favorire l'attrazione di nuovi investimenti produttivi in attività innovative dall'Italia e dal mondo. L'auspicata riforma del fisco deve costituire in termini metaforici un'autentica rivoluzione copernicana soprattutto nei rapporti tra amministrazione finanziaria, cittadini ed imprese, perché, pur essendo importante riformare gli aspetti tecnico-economici del sistema (dal complesso al semplice, dalle persone alle cose, come ama dire il Ministro dell'economia), se non si risolve alla radice l'evasione fiscale, che insieme alla bassa crescita è la vera piaga italiana, il sistema resterà sempre malato e sempre in affanno. Per quanto riguarda le scelte in tema di energia, il ritorno al nucleare è indubbiamente una scelta che si impone per ragioni legate al soddisfacimento del fabbisogno del Paese di sicurezza energetica e di competitività del sistema produttivo. Non bisogna però dimenticare che nelle concrete scelte, soprattutto quelle riguardanti la localizzazione degli impianti e lo stoccaggio delle scorie, le comunità locali dovranno essere parte attiva nel processo decisionale. La giusta importanza va poi riconosciuta anche agli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile e al risparmio energetico, soprattutto in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di un'economia rispettosa dell'ambiente. Non bisogna dimenticare poi, come ricordavano i relatori, le politiche della concorrenza e della liberalizzazione da perseguire senza esitazione in diversi comparti dell'economia nazionale, compreso quello dei servizi professionali, alle quali però il documento riserva uno spazio ancora insufficiente, senza prefigurare precisi impegni circa le misure concrete da attuare. Infine, vogliamo richiamare l'attenzione del Governo sull'urgenza di imprimere una svolta alla questione lavoro. Non sono soltanto i dati sulla crescente disoccupazione a preoccuparci (quella giovanile al Sud è arrivata a livelli intollerabili per un Paese civile); ci preoccupa anche la generale condizione di precarietà, di instabilità e di incertezza che avvolge tutto il mondo del lavoro in Italia, dove proprio i giovani, sui quali si dovrebbe investire di più in termini di formazione del capitale umano per assicurare al Paese lavoro di qualità in futuro, sono i più penalizzati, costretti a lavori precari e temporanei presso imprese che proprio per questo non trovano utile investire su di loro. Pensiamo che dare soluzione alla questione lavoro sia una condizione fondamentale, oltre che un primo importante passo verso la ricostruzione di una economia e di una società che pongono al centro l'uomo, il suo lavoro, le sue aspettative e i suoi diritti. È questa la pietra angolare della società che vogliamo. Ciò detto, Futuro e Libertà per l'Italia dichiara il proprio voto favorevole.

Grazie,

sottoscrivo in pieno le sue considerazioni, sia quelle critiche rispetto al documento della maggioranza, sia quelle propositive che si traducono nella risoluzione presentata. che risponde ad una precisa domanda: colleghi, tornano i conti? Sappiamo che in queste ore il Ministro dell'economia sta svolgendo un serrata verifica sulle risorse

dall'università (riforma che quest'Aula ha varato), alle politiche per le missioni internazionali, agli ammortizzatori sociali e agli altri interventi di cui si discute.

è necessario sottolineare, senza polemiche inutili, ma con una constatazione obiettiva, che in questi ultimi due anni e mezzo la spesa è salita,

che complessivamente tutti i tagli che si propongono al bilancio dello Stato si infrangono oggi con i ritardi nella definizione dei costi standard, e dunque di un approccio di un approccio virtuoso in materia di contenimento della spesa territoriale. Oggi si apre la Conferenza dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani in cui si ricorda che i Comuni hanno fatto il proprio dovere e si trovano con riduzioni drammatiche dei bilanci degli enti locali; ma, alla fine, nel nostro Paese i numeri fondamentali sono questi: cresce la spesa al netto degli interessi e cresce in particolare sui livelli regionali. La conclusione è quella che indubbiamente ha visto oggi una larga concordanza di principio in quest'Aula. L'unica soluzione non è certo quella di aumentare le tasse, né quella di affrontare ulteriori salassi impossibili per la spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio è stato contestato ieri in due luoghi in cui non può far tornare i conti.

in cui le difficoltà per la ricostruzione dell'Aquila, come era stato promesso, sono davanti agli occhi di tutti gli italiani. La coperta è corta, le promesse non possono essere realizzate. La conclusione è quella contenuta, come documento di indirizzo, nella mozione da noi presentata, ovvero in coraggiose politiche per il ritorno alla crescita. Se non si produce più ricchezza, da dove si prendono i soldi, posto che non si può ulteriormente comprimere la spesa

È evidente che lo si può fare con coraggiose politiche per la crescita. Questo è lo sforzo che si evince nel terzo documento che si voterà. È chiaro che una mozione parlamentare

contenendo con ogni probabilità, rispetto ai 7 miliardi che dovranno essere messi in campo, un'indicazione generale che poi dovrà essere tradotta in norme.

Azzollini ci sta lavorando - più ampia che non quella dei firmatari dell'attuale mozione: una convergenza larga del Parlamento sulle tematiche della crescita economica.

campo, guardando al futuro politico, oggi così incerto, della maggioranza e dell'orizzonte politico-parlamentare del nostro Paese, che, se su qualcosa bisogna unirsi,

di adottare quelle misure per la crescita economica che siano in grado di dare una scossa al nostro Paese.

è stato svolto in tre successive circostanze ed ora ci accingiamo a votare), il senso di questo documento, con i suoi limiti - di cui mi scuso - e con le sue potenzialità, che non sono del tutto insignificanti, è proprio quello di indicare

che non è di Bondi la colpa del crollo di un edificio nella

fatto che è caduto l'alibi dell'Europa. Infatti, fino a quando si dovevano affrontare scelte impopolari e difficili, effettuando tagli drastici e draconiani, allora vi era l'alibi dell'Europa; oggi che l'Europa ci chiede di fare molto di più di quanto il Governo e la maggioranza stanno portando avanti, si fa finta che non si riescano a capire

non solo con la contrattazione decentrata di secondo livello, non solo con la la sicurezza sul lavoro (detto poi da un Governo e da una maggioranza che sono andati avanti con proroghe e proroghe delle misure a sostegno della sicurezza del lavoro),

l'Europa ci sta chiedendo - e sta chiedendo agli Stati membri - di concordare delle politiche economiche da portare avanti nei prossimi mesi del nuovo anno.

che è un atto formale. È stata presentata dal Ministro dell'economia come un atto formale, che si limiterà semplicemente ad alcune tabelle finanziarie in cui verranno

non possiamo considerare questo documento come un atto puramente formale o una semplice bozza. L'Europa ci dice chiaramente di individuare gli obiettivi di politica economica nazionale e le misure conseguenti da adottare: una coerenza, una compatibilità anche economica con gli annunci che si fanno. Questo documento altri lo hanno definito un «copia e incolla», un atto burocratico che è la sommatoria di piccole relazioni dei Ministeri. In realtà non è altro che un semplice collegamento tra ciò che non si è fatto prima e ciò che non si è in grado,

nel merito, alcune considerazioni molto semplici. Nella nota introduttiva a questo Programma nazionale di riforma (che è poi l'impianto di tutto il Programma) si scrive si scrive che nella strategia di sviluppo del nostro Paese vi è un vincolo e vi sono quattro obiettivi. Il vincolo è dato dal debito pubblico, e, detto da una maggioranza e da un Governo che in un anno lo hanno aumentato di 150 miliardi di euro, è detto tutto.

in un compartimento stagno e far finta di ignorare cosa sta accadendo in queste ore nell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco al fatto che una legge di stabilità, di stabilità, presentata come elemento e leggero innovativo, è stata bloccata dal Ministro dell'economia per problemi interni alla maggioranza, perché il Governo è andato sotto

nel cosiddetto decretino per lo sviluppo, in cui si stanno cercando risorse, e una risorsa importante per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese il pacchetto giochi: si potenzierà il sistema del *poker on line*. Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non funziona, che, accanto a questo galleggiamento, l'altro ostacolo alla crescita ed allo sviluppo del nostro Paese è l'assenza di credibilità di questa maggioranza. Il senatore Morando poc'anzi ha richiamato l'attenzione dell'Aula sul *trend* di crescita che stanno avendo la collocazione e la vendita dei titoli di Stato del nostro Paese. Dobbiamo collocare nei prossimi mesi 44 miliardi di euro tra BOT e CCT e quello che l'agenzia di *rating* Standard & Poor's ha messo in risalto è che questa collocazione sarà estremamente difficile, per via della perdita di credibilità e della instabilità politica che si sta creando nel nostro Paese. Ci rendiamo conto, signor Presidente, che alcuni analisti economici internazionali, di fronte alla collocazione di un pacchetto di Buoni del tesoro poliennali con un aumento degli interessi dal 3,90 al 4,01, hanno incominciato a parlare

parlando di zone a burocrazia zero o di fiscalità di vantaggio, che è una pura chimera, con l'abolizione di IRPEF e l'IRAP, che le Regioni del Sud non possono attuare; equità fiscale e di riforma fiscale, facendo credere che i decreti legislativi attuativi del federalismo possano risolvere il problema, quando sono soltanto sulla carta e stanno avendo un'accelerazione solo mediatica;

invito i senatori della maggioranza ad affrontare la questione legale come consiglia

Signor Presidente, è proprio difficile non essere d'accordo su quanto è scritto in questo progetto di Programma. Era anche difficile non essere d'accordo, verso la fine degli anni Ottanta, con un personaggio televisivo che compariva in una trasmissione di successo; si chiamava Catalano e diceva cose molto ovvie, tipo: «è meglio invecchiare ricchi e in buona salute che non poveri e malconci». Questo mi pare il tema

con una fiscalità più giusta. Quel che manca, a mio avviso, è l'elemento fondamentale, ovvero l'intelligenza politica. Sono due gli attributi della intelligenza umana: umana: la capacità di sintesi e la capacità di adattamento. In politica, io credo che l'attributo sia la capacità di individuare strumenti e individuare delle priorità. In questo documento difettano gli strumenti ed è assente la priorità. Già ieri, nella discussione in 7a Commissione, esponente della maggioranza, con atteggiamento intellettualmente onesto, faceva notare questa difficoltà e questo imbarazzo. Ancora questa mattina, in alcuni passaggi, sempre un autorevole esponente della maggioranza diceva che il Governo ha forse difficoltà perfino a capire quale sia l'entità del vincolo:

Ebbene, in assenza di questo atteggiamento vero della politica, che assuma su di sé la capacità di indicare la strada e le priorità e di dare sviluppo concreto a degli strumenti, mi pare proprio difficile dire che siamo di fronte a un documento di respiro. di respiro. Noi non usciremo da questa vicenda se non individuiamo al più presto una priorità vera, alla quale indirizzare le risorse che devono essere prese dove è possibile e consentito prenderle.

una proposta autenticamente pragmatica, sia una strada. Però, sul tema delle priorità, mi sia consentito davvero sottolinearne una: e speriamo che non sia soltanto un ritornello. Quando, alla fine degli anni 80, sempre dopo la caduta del Muro di Berlino, la Germania assunse la straordinaria sfida dell'unificazione unendo a quel Paese federale un Paese che aveva difficoltà a produrre, difficoltà ad avere ricchezza, difficoltà anche in termini di corruzione e di criminalità, quella classe dirigente fece una scelta sopra tutte le altre. Tale scelta è scritta, è deliberata ed è storicamente significativa: prese i migliori insegnanti della Germania occidentale, li mise in condizione di essere riconosciuti come elemento fondamentale della società e li mandò a insegnare nella Germania orientale. Insomma, investì sulla scuola, investì sulla formazione e investì sull'università: i risultati, dopo 20 anni, possono vedersi.

Questo creerà una disaffezione nei confronti di un Paese che non sa formare i propri figli e finirà con il creare una situazione di lontananza dei cittadini dal Paese. Se noi non interveniamo in tempo in questo settore, avremo una gravissima responsabilità nell'aver creato una cittadinanza meno vincolata ai destini della propria nazione. Io credo che di questo si parli quando ci si accinge a immaginare il proprio Paese nei prossimi dieci anni (e forse qualcosa di più): la capacità di un sogno che si concretizza in un progetto e che diventa un programma. Non può essere tutto insieme. Nel documento del Governo il sogno si confonde con il progetto e il progetto con il programma; occorre invece avere chiarezza di percorso per consentire che la pragmaticità, che la politica deve declinare, sia una realtà. Per questo ci pare di poter cogliere con qualche difficoltà la proposta di risoluzione della maggioranza; ci pare di poter dire che, forse, ragionando intorno ad alcuni elementi condivisibili della mozione del senatore Rutelli, si possa fare un passo

e documenti sarebbero stati il Programma nazionale di riforma e la legge di stabilità. Con puntualità, arriviamo a discutere di questo argomento,

discusso nel famoso semestre europeo. Non siamo qui per un mero dovere di norma relativamente a delle scadenze, ma per una convinzione e un impegno forte, fattivo, efficiente ed efficace nel contrastare la crisi economica che ha colpito non solo l'Europa, ma tutto il mondo; per dare stabilità e sicurezza alle nostre famiglie e alle nostre imprese e per vedere con più positività un futuro che dà segnali incoraggianti, che devono essere sostenuti. il Governo in questi giorni vanno in tale direzione. Non dobbiamo dimenticarci, parlando di scenario europeo e del bisogno di una *governance* integrata,

sui titoli e sui *bond*. Si tratta di un fatto assolutamente normale, vivendo in un sistema europeo con una moneta ormai unica. È quindi assolutamente ridicolo

di *gossip* assolutamente estranee a queste dinamiche. L'hanno fatto anche autorevoli persone; sembra veramente che ci sia, ne sono convinto, una strumentalizzazione che fa assolutamente male al Paese e che non è assolutamente collegata con i dati di fatto.

votato una coalizione e un Governo delle persone: il popolo deve decidere, la potestà è dei cittadini e degli elettori; con intrighi di palazzo, pensare di ribaltare la volontà popolare. Quindi non ci riconosciamo in queste affermazioni del collega Morando, pur apprezzando alcune analisi economiche, assolutamente condivisibili. sono il passaggio obbligato, non solo perché lo crediamo fortissimamente e lo testimoniamo con questo documento, ma anche

e che non è stata toccata dalla crisi economica come gli altri Paesi che prima ho citato. Stiamo vedendo anche le forti azioni che sta mettendo in atto il nuovo Governo inglese, con manovre finanziarie fortissime

ringrazio - con una manovra, il famoso decreto-legge n. 78, che ha continuato una riforma che era negli anni, dando garanzia e sicurezza ai conti pensionistici rispetto al PIL di questo Paese. Un'altra grande misura

siamo forse ancora indietro. Abbiamo un esempio virtuoso, rappresentato dalla Germania; in particolare ho ricordato in quella discussione i contratti Volkswagen o i contratti regionali, che auspichiamo e sosteniamo da tempo.

ricordando che con il federalismo, che è un processo di riforma strutturale del nostro Paese che partirà in maniera forte dal 2012 e si completerà nel 2014,

e credo che sia giusto da parte dell'opposizione, della principale forza dell'opposizione, il Partito Democratico, rivendicare di avere voluto che il Parlamento se ne accorgesse, si accorgesse che stavamo, vivendo un passaggio storico con l'approvazione di questo nuovo modello di *governance* economica europea da parte del Consiglio europeo

accanto all'altro che dovrà rapidamente avvenire, quello sul piano di stabilità. Credo non sia esagerato definirlo un passaggio storico e, tuttavia, signor Presidente, questo non si direbbe direbbe - come veniva detto anche dai colleghi della maggioranza - sfogliando la stampa, i *media* del nostro Paese, che sono in ben altre faccende affaccendati e appassionati;

del Presidente del Consiglio. È stato ricordato stamattina come tutti i Capi di Governo abbiano posto in cima alla loro agenda il confronto su questi temi: tutti i Capi di Governo europei tranne il nostro Presidente del Consiglio,

Il nostro Presidente del Consiglio, invece, non ha proferito verbo su questa questione, e non abbiamo avuto il dono di vederlo in Parlamento. E non abbiamo visto in Parlamento neppure il ministro Tremonti, che pure è stato il *dominus* di questo *dossier*: lui, che ha fatto parte della *task force* e che ha partecipato al confronto in sede di gruppo di lavoro a Bruxelles e che, quindi, ha predisposto gli atti e partecipato a nome dell'Italia all'elaborazione del Piano. Non abbiamo visto il ministro Ronchi, che pure è il primo firmatario del programma di riforme: non si è presentato. E non E non abbiamo avuto il dono di un confronto con il ministro Frattini sulle implicazioni di politica estera che questo passaggio storico comporta per l'Europa e per il nostro Paese. Insomma, signor Presidente, così non va, e noi le chiediamo, anche in qualità di Presidente del Senato, di far osservare al Governo questo aspetto. Se non fosse stato per l'opposizione, il Parlamento sarebbe stato completamente bypassato in questo passaggio storico per l'Europa e per il nostro Paese. Perché sia un passaggio storico per l'Europa è stato detto ampiamente e, quindi, non lo ripeto; ma in sostanza c'è un capovolgimento nella procedura di governo delle politiche economiche, nel rapporto tra gli Stati e l'Unione, con una significativa - verrebbe da dire spettacolare - cessione di sovranità da parte degli Stati nei confronti dell'Unione. un fatto che salutiamo come enormemente positivo, perché abbiamo detto per anni che accanto all'unione monetaria ci doveva essere una gamba dell'Unione sulle politiche di bilancio ed economiche. Finalmente questa gamba c'è;

il merito di queste politiche economiche che vengono scelte e decise a livello europeo. Siamo assolutamente d'accordo con il rigore: non ci può essere crescita se non c'è rigore, e il collega Morando, oggi, ha spiegato benissimo come il debito, non solo non sia stato fatto per sostenere la crescita, ma sia oggi uno degli elementi che più impediscono la crescita delle economie europee, in particolare di quelle indebitate come la nostra. Ma, accanto al rigore, ci deve essere la politica di espansione, la politica di investimenti da parte dell'Unione, non solo dei singoli Stati, valorizzando al meglio quella risorsa inestimabile che è la nostra moneta comune.

per cercare di unificare le forze politiche del nostro Paese nel chiedere in maniera impegnativa in Europa una politica di investimenti fondata sugli euro-bond, euro-bond, utilizzando quindi al meglio la forza della nostra moneta. Non si capisce perché il Governo non ne abbia fatto una posizione negoziale forte, determinata, precisa e convinta.

costruire gli strumenti per una politica di investimenti a livello europeo. L'altro grande tema è quello della sovranità politica e della democrazia. La Lega per anni ha posto questo problema: la democrazia che si interrompe nella tecnocratica Bruxelles. È un tema che ha un suo fondamento, anche se è stato agitato in modo propagandistico e dal nostro punto di vista inaccettabile. Tuttavia proprio questa era l'occasione per

è, anzitutto, quale sia la prospettiva. Pensiamo che la prospettiva debba essere quella della costruzione di una vera unione politica, dopo avere costruito - e la stiamo costruendo sempre più - l'Unione economica. Pensiamo vi debba essere quanto prima da parte dei popoli europei l'elezione di un Presidente degli Stati Uniti d'Europa, che possa essere il titolare primo di una politica economica e delle grandi scelte che riguardano il destino di tutti i popoli d'Europa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore in una fase intermedia che probabilmente sarà lunga, diventa cruciale il rapporto tra Parlamenti, opinioni pubbliche nazionali e Governi, perché se le decisioni le prendono i Governi è essenziale che queste siano legittimate democraticamente presso le rispettive le rispettive opinioni pubbliche. Oggi ciò non avviene, in modo particolare nel nostro Paese, come dimostrano i banchi del Governo che sono rimasti sistematicamente vuoti, almeno nei livelli delle massime responsabilità, dall'inizio alla fine di questo percorso. Se il rapporto tra Governo e Parlamento è opaco, ciò costituisce non solo una ferita che viene inferta al corpo del Parlamento, ma un disastro dal punto di vista della costruzione del consenso attorno a politiche impegnative. Abbiamo davanti a noi da scalare, come dirò brevemente: come possiamo pensare di farlo senza preparare a questo il Paese, senza parlare di questo con il Paese, con le forze sociali e l'opinione pubblica? Il Paese deve essere pronto ad affrontare un passaggio così difficile e delicato, altrimenti come faremo nei prossimi mesi a rendere possibili le decisioni impegnative che dobbiamo affrontare? Ed ecco allora il terzo ed ultimo punto. Questo è un passaggio storico per l'Italia,

un Programma di risanamento. Riforme e risanamento che sono la scalata di una parete di sesto grado. Noi, come è stato già detto, debito probabilmente dovremo trovare qualcosa che si avvicina ai 40 miliardi di euro nei prossimi cinque mesi, perché è entro aprile che va presentata una manovra del genere. Il Paese questo non lo sa, e non lo sa perché non c'è un Governo che glielo dica. Allora, è evidente che non potremo affrontare un passaggio di questo genere con una incertezza, una precarietà, una instabilità politica come quella che abbiamo davanti a noi. Oggi il senatore Grillo ha detto che solo il centrodestra è in grado di fare una manovra che consenta di stare dentro i vincoli europei. Benissimo, fatelo. Avete i numeri per farlo. Di fronte alla crisi che il Paese sta vivendo, di fronte alla drammatica crisi politica che il Paese sta vivendo, se il centrodestra è in grado, se voi siete in grado di dare ancora un governo al nostro fatelo nelle prossime ore: non c'è più tempo da perdere. Se non siete in grado di farlo, andate dal Presidente della Repubblica e consegnate a lui la responsabilità di trovare un percorso nuovo per il Paese. Un percorso che consenta all'Italia di affrontare il passaggio storico nel quale siamo immersi

Signor Presidente, sarò molto breve, anche perché fra non molto dovremo riformulare la mozione presentata dal senatore Rutelli, che ci impegnerà qualche attimo, sempre su questi temi. Mi soffermo soltanto su due rapide questioni. La prima è metodologica. Voglio dire con un pizzico di orgoglio che in Senato continuiamo a scrivere delle belle pagine parlamentari, signor Presidente. La La mozione che abbiamo votato la scorsa settimana sulle questioni dell'Unione europea, sulla revisione del Patto di stabilità e crescita e della *governance* macroeconomica della Commissione europea

il senatore Massimo Garavaglia, ha potuto produrre un documento che ha un significato particolare, perché espresso dal Senato nel suo complesso, quindi con la fattiva collaborazione ed anzi costitutiva collaborazione anche dei colleghi dell'opposizione.

oggi è il 10 novembre, e anche in questo caso, grazie anche a un'intesa politica tra i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione, abbiamo potuto fare una discussione, che si chiuderà magari questa volta con un voto diverso. È ovvio, infatti, che la maggioranza sin d'ora a mio nome mio nome approva il Programma di riforma che il Governo presenterà il 12 novembre in sede europea e che i colleghi dell'opposizione invece mantengano, ovviamente, le loro differenze, ma il Senato della Repubblica, il Parlamento si è occupato di questo: è stato all'altezza del dibattito in tutta Europa ed ha connotato in questo momento l'Italia come una delle Nazioni che, insieme con le altre, con il suo Parlamento dà delle indicazioni precise in seno all'Unione europea. È qualcosa che in questi giorni non ha molto successo sui *media,* ma che invece ha successo in queste Aule e, a mio avviso, tutti insieme, sotto questo profilo, scriviamo una pagina parlamentare degna di nota. Questo è secondo me l'elemento più significativo del dibattito. All'interno di ciò naturalmente sia la precedente discussione, sia quella in corso hanno presentato una varietà di opinioni, ma anche una convergenza su alcuni temi che mi paiono assolutamente rimarchevoli.

è necessario concentrare l'azione del Governo e del Parlamento nella seconda metà della legislatura su riforme e provvedimenti mirati alla promozione della crescita economica, impegna il Governo a promuovere iniziative di competenza al fine di realizzare i seguenti obiettivi, che concorreranno a formare l'agenda per la crescita, nonché il Programma nazionale di riforma per la Strategia europea «per l'occupazione ed una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» nel decennio 2010-2020: migliorare i servizi e le prestazioni sociali per i cittadini riducendo la spesa pubblica e bloccando l'espansionismo delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali. In particolare, va va operata la riduzione dei costi della politica, va operata la revisione dei meccanismi di spesa dello Stato ma non sulla base di tagli lineari, che spesso provocano impatti negativi, iniquità e inefficienze, come nei comparti della cultura e della scuola. effettuato il taglio dei margini di spreco e inefficienza nella sanità mediante accorpamento delle Aziende sanitarie locali centralizzazione degli acquisti, ridefinizione dei fabbisogni sovradimensionati. Il federalismo deve essere anche competizione tra le istituzioni pubbliche perché la certezza di adeguate ed eque prestazioni per tutti i cittadini nei campi della salute, dell'istruzione e formazione e dei servizi sia anche frutto dell'esercizio di parametri concorrenziali che consentano agli utenti di scegliere i servizi migliori e comportino premi per le prestazioni più efficaci. migliorare la competitività del sistema-Italia, tenendo conto che l'accelerazione delle riforme è parte di uno sforzo strategico coordinato per accrescere la competitività del Paese rispetto alle sfide dell'economia globale: è con riforme e competitività che si dà la migliore risposta alla «questione settentrionale». La svolta per la «questione meridionale» va trovata con certezza di risorse, spendendo quelle disponibili, finora in parte inutilizzate, per realizzare i progetti che attivino investimenti pubblici, privati ed europei e porre nel prossimo decennio il nostro Mezzogiorno - anche creando zone franche economiche - al centro della crescita del Mediterraneo. La «questione giovanile» - alta disoccupazione, blocco dell'ascensore sociale, sfiducia diffusa - è diventata una drammatica questione generazionale, e non si risolve affatto con provvedimenti settoriali o assistenziali, ma con un'economia più aperta che accresca le opportunità, con particolare attenzione alla riorganizzazione delle professioni ed alla formazione. Va consolidato e innovato il nostro ancoraggio europeo a partire dalle possibilità di sviluppo che scaturiranno dai nuovi settori del Mercato unico. Le liberalizzazioni rimangono urgenti e vanno ulteriormente tradotte in disposizioni legislative; vanno rafforzate le norme in materia di servizi pubblici locali per evitare la spinta verso l'alto delle tariffe. È tempo di avviare la stagione delle riforme della giustizia nell'interesse del cittadino, sia sul piano del processo civile che sul piano del processo penale, anche attraverso l'eventuale ricorso ad organismi individuati dal Parlamento.

futuro Ministro dello sviluppo economico sarà chiamato a coordinare le azioni prioritarie per i nostri comparti manifatturieri - che con le esportazioni oggi sorreggono la pur debole crescita del PIL - promuovendo le capacità del *made in Italy*, le produzioni di qualità, il settore energetico e i comparti innovativi. Non c'è progresso senza miglioramento della scuola, dell'educazione, della conoscenza: c'è bisogno di una stagione di buone direttive, investimenti in innovazione e buona amministrazione. degli enti territoriali; *n)* l'economia verde ha grandi potenzialità nei settori della logistica e dei trasporti, dell'efficienza energetica nell'edilizia, delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili. La concentrazione di questi fattori - indispensabili per centrare gli obiettivi vincolanti concordati in sede europea, e per la conquista di nuovi mercati - riguarda fortemente le città, motori dello sviluppo sostenibile. Ma occorre che la regolazione sia resa chiara, semplice, e soprattutto omogenea. L'Italia deve porsi all'avanguardia per migliorare l'ambiente e conquistare i mercati che si apriranno con la direttiva 2010/31/UE, che imporrà nell'arco di un decennio la costruzione di edilizia a zero emissioni; La competitività da ritrovare e la coesione nazionale dipendono da vari fattori principali: 1) il contrasto della corruzione; 2) la crescita della produttività, che è anche condizione per attrarre investimenti esteri, e modelli contrattuali che sviluppino la contrattazione decentrata di secondo livello e coinvolgano i lavoratori nei risultati dell'impresa; l'effettiva premialità per la responsabilità e il merito anche nelle amministrazioni pubbliche; un nuovo codice del lavoro semplificato, anche sulla base delle proposte del disegno di legge n. 1873; 3) un nuovo ordine liberale e il tessuto civile dell'economia. In proposito, occorre tener conto che: le relazioni tra le persone, l'intraprendenza diffusa e il ruolo delle famiglie sono stati gli assi portanti delle stagioni d'oro della crescita italiana.

ad accogliere le proposte di riformulazione che il collega Azzollini ha fatto, però preannuncio che chiederò di mantenere due votazioni: quella sul testo della mozione come riformulata e

Presidente, la mozione è stata pressoché riscritta nella sua articolazione attraverso l'espunzione di parti anche importanti e la modifica di altre. che il senatore Rutelli ha appena chiesto la votazione comunque di quelle parti non accolte dalla maggioranza, sulle quali quindi ci dovremo esprimere. Bisognerà vedere anche come queste si collocheranno rispetto al testo che è stato riformulato dal presidente Azzollini. Per queste ragioni, tenendo conto della complessità

Presidente, è evidente che la richiesta di maggior approfondimento, dal mio punto di vista, non può che essere rispettata e in principio accolta.

Signor Presidente, come Italia dei Valori non abbiamo nulla in contrario, anzi assecondiamo la proposta del Partito Democratico di avere un po' di tempo a disposizione per per approfondire la riformulazione della mozione Rutelli. Per quanto riguarda, invece, la proposta del senatore Rutelli di procedere

comunque che avvengano più votazioni sulla base dei capoversi stralciati. Ciò, in quanto vi sono alcuni aspetti che hanno il nostro assenso e altri no.

nell'*iter* che ha avuto la mozione presentata dal senatore Rutelli. Questa mozione è stata presentata da diverse settimane. Come ben sa il senatore Rutelli e come sanno i Capigruppo di tutti i Gruppi,

la necessità di discuterla dopo che si erano esauriti altri punti all'ordine del giorno, e la mozione è stata rimessa all'ordine del giorno su mia proposta, prima ancora che tutti i Capigruppo, compreso il presidente del Gruppo del senatore Rutelli, ovviamente condividessero. Abbiamo mantenuto come maggioranza - non solo il mio Gruppo - la massima attenzione e ci siamo confrontati (il senatore Azzollini è il presidente della Commissione bilancio, non un passante) ritenendo di esprimere la nostra proposta di cosa condividevamo e cosa no. Le mozioni vengono presentate per trovare condivisione. Se il senatore Rutelli su alcune parti ha accettato una riformulazione, noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni per procedere al voto. In caso diverso, se il senatore Rutelli, ho ascoltato l'intervento, ritiene che si debba procedere diversamente, andremo avanti con il calendario che è stato fissato e ridiscuteremo la questione in un'altra fase dei lavori del Senato, quando la Conferenza dei Capigruppo fisserà nuovamente questo tema. Su questo vorrei essere molto chiaro, alla luce della mia richiesta di discutere, come mi ero impegnato a fare, questa mozione, il senatore Rutelli lo sa benissimo. Quindi, o si vota ora, oppure, se il senatore Rutelli, che è titolare della mozione, lo ritiene, fisseremo un'altra discussione sulla riformulazione della mozione e su quant'altro. Questo vorrei che fosse molto chiaro, e lo dico perché sono stato io a ricordare che in Aula bisognava portare la mozione del senatore Rutelli.

abbiate, superannotato, che dovrebbe descrivere qual è il contenuto della mozione, ma quello l'ho ascoltato dalla voce del senatore Azzollini e quindi, sia pure

quali sarebbero le parti che non sono da ritenersi accolte, perché tra quelle accolte ci sono riformulazioni del testo originario. Mi chiedo se le parti non accolte sono anche quelle che sono rimaste fuori dalla riformulazione oppure sono parti che non sono in alcun modo rientrate nella riformulazione. Faccio un esempio per tutti:

Dopo aver votato in qualunque modo il testo Azzollini? E potrei continuare. Potrei anche chiedere: poiché nella versione che è stata letta dal presidente Azzollini

organismi individuati dal Parlamento, posso interloquire su questa riformulazione e chiedere che questa parte venga espunta? È cioè quello che lei, poco fa, non ha detto, presidente Schifani, perché è un presidente come si deve, che si esprime correttamente, e che non posso dire io, perché sono presidente di un Gruppo parlamentare, ma che in un «conversario» privato probabilmente ci diremmo.

innanzitutto, il mio *incipit* sull'inizio di questo tipo di votazione relativa alla mozione lasciava trasparire, ovviamente, da parte della Presidenza, non un imbarazzo, perché noi siamo qui per onorare il nostro ruolo, ma sicuramente il pericolo che l'Aula non fosse compiutamente messa in condizione di capire e sapere quello che stava votando. Siccome dovere della Presidenza è quello di mettere l'Assemblea - ogni singolo senatore - in condizione di ben comprendere, leggere e sapere quello che sta votando, la mia preoccupazione è trasparita immediatamente dalla mia battuta, che era ampiamente serena. Non vi è dubbio, tra l'altro, che le osservazioni della presidente Finocchiaro siano pertinenti perché, in questa mozione, quando vi sono delle integrazioni su alcuni principi, votate le integrazioni precludono, invece, quelle parti alle quali si sovrappongono perché esprimono un principio diverso. Un conto, infatti, è dire che si riforma la giustizia ricorrendo a una composizione parlamentare fatta da magistrati, avvocati e 15 parlamentari, con questo organismo; altro conto è riformare la giustizia attraverso, eventualmente, organismi *ad hoc*. Se si approva questa seconda parte, non vi è dubbio che la prima sia preclusa. Allora, perché rimetterla in votazione? Colleghi, passo

quali parti vengono precluse dal contesto generale perché contraddittorie.

la pregherei di considerare l'ipotesi di espungere quelle tre righe in quel capoverso, perché mi sembra che si potrebbe dar luogo ad una votazione contraddittoria del Senato sullo stesso argomento nel corso della stessa discussione, sia pure trattandosi di due strumenti diversi. sostanzialmente peccheremmo di ripetitività, ma non è che ci contraddiremmo. MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, purtroppo mi permetta di far notare che non è così, perché la risoluzione sul Programma nazionale di riforma contiene proposte al Governo, per la sua integrazione, diverse da quelle che contiene questa mozione.